Onorevoli colleghi, ricorre oggi il 7° anniversario del terremoto che nel 2009 colpì L'Aquila e altri 57 Comuni abruzzesi causando 309 vittime e migliaia di feriti e sfollati. Il cratere che nella notte del 6 aprile si è aperto nel centro storico dell'Aquila è la fotografia, impressa nella mia e nella memoria di tutti gli italiani, della portata distruttiva di quel sisma che in pochi minuti ha spezzato centinaia di vite e inghiottito una parte della storia di una città. A questo personale e doloroso ricordo si accompagna però la memoria di una incredibile solidarietà dimostrata

è un modo concreto per non dimenticare quel momento, quel sisma. Ma per tornare alla normalità abbiamo il compito di restituire pienamente al tessuto cittadino e sociale aquilano la propria identità. solo conservando con orgoglio la propria storia che il popolo abruzzese potrà guardare alla ricostruzione con speranza. Come ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella il 16 novembre scorso in occasione della visita alla città, «L'Aquila si appresta a vincere questa difficile prova, portando la propria identità e la propria storia in un domani migliore». Con questo auspicio, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 ed esprimo tutta la mia personale vicinanza, insieme a quella di tutta l'Aula, a tutto il popolo abruzzese.

Signor Presidente, proviamo un dolore fortissimo, un dolore che probabilmente non andrà mai via dal cuore di tutti gli italiani, come ha detto lei prima. In concomitanza con la ricorrenza del tragico 6 aprile, si riapre dentro di noi una ferita enorme, che resterà sempre aperta, anche quando sarà stata ultimata la ricostruzione. L'Aquila, infatti, non è solo un capoluogo, ma è un simbolo, ma è un simbolo, una comunità operosa, una città con un patrimonio architettonico veramente importante, non solo per la Regione Abruzzo, ma per l'Italia intera. Prima si ricordavano i numeri drammatici di quella tragedia i danni subiti. Sono i numeri del terremoto che il 6 aprile del 2009 ha colpito l'Aquila e i comuni vicini. Numeri imponenti, che non bastano però per descrivere il reale significato che ha avuto la catastrofe per l'Abruzzo e per il nostro Paese. Il sisma infatti ha distrutto una delle più belle città medioevali d'Italia, ha colpito una delle più grandi e vitali università del Centro-Sud, creato un caso scientifico internazionale e portato a galla l'ennesimo esempio del malaffare e corruzione nel nostro Paese. Una ferita vecchia ormai di sei anni, ma che per certi versi stenta ancora a rimarginarsi. Oggi siamo qui a ricordare, oggi siamo qui per non dimenticare, siamo qui per chiedere una soluzione ed una risposta alle tante domande finora inevase. Pochi mesi fa questa Assemblea ha votato favorevolmente alla richiesta di costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta. Ci auguriamo che finalmente la verità possa emergere e auspichiamo soprattutto che possa essere fatta giustizia per i cittadini e per le imprese dell'Aquila e degli altri paesi colpiti,

resta una città gentrificata dai suoi quartieri nuovi. A proposito, sono quasi stucchevoli le discussioni sulla qualità dell'edilizia della *new town*, quando invece il dato più drammatico è che lì si sono realizzati rioni e quartieri dormitorio, dove il sistema delle relazioni sociali è stato annientato. Sembra un paradosso, ma nel 2016, a fronte del recupero di moltissimi centri storici da parte dei piccoli e grandi comuni italiani, dobbiamo registrare che lo Stato (dopo ben quattro Governi) ancora non riesce a ricostruire L'Aquila. I lavori sono perennemente in corso, la vergogna cresce!

309 vittime, migliaia di feriti, distruzione del centro storico e di interi quartieri della città capoluogo della Regione Abruzzo e di 57 Paesi della provincia, il cratere, con migliaia di sfollati. Simbolo e memoria di quel sisma furono i tanti giovani morti, ospitati nella Casa dello studente, dove una parte della palazzina crollò sbriciolandosi; di cui 50 universitari cosiddetti "fuori sede" molti dei quali si trovavano quella notte all'Aquila, perché nei giorni seguenti avevano lezioni ed esami. Purtroppo di quell'evento si ricordano anche i pensieri e i ragionamenti di sciacalli, che, a distanza di poche ore, già pensavano agli affari della ricostruzione, cosa che ha fatto aggiungere rabbia al forte dolore. Anche quest'anno, come nei precedenti anniversari del terremoto, si è svolta, con rinnovata commozione, la fiaccolata commemorativa che si ripete da sei anni e che è culminata, in piazza Duomo, con la lettura dei nomi delle 309 vittime. Quello dell'Aquila è uno dei tanti eventi di calamità naturale che nel corso della storia, anche la più recente, hanno colpito il nostro Paese. Purtroppo, però, anche in questo *post* terremoto si sono manifestate opacità, malagestione delle risorse (vorrei ricordare che sono già stati spesi 11 miliardi e che altri 7 se ne aggiungeranno), irregolarità, illegalità, lentezza nella ricostruzione e problemi, soprattutto nell'edilizia scolastica. Per i cittadini dell'Aquila e dei paesi del cratere, soprattutto per i parenti alle vittime, che si sono costituiti in associazione,

proseguire l'*iter* per la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione, per portare alla luce le patologie emerse sia nell'emergenza, sia durante la ricostruzione. Il Gruppo parlamentare della Lega Nord Autonomie esprime sentimenti di cordoglio a tutti i familiari delle vittime e di vicinanza al popolo aquilano ed assicura il massimo impegno per contribuire a rimarginare le profonde ferite che la tragedia del 6 aprile del 2009 ha provocato.

continua in questi giorni. Il fatto che ci siano 424 cantieri oggi aperti è molto significativo.

per i terremotati (le *new town*), alloggi che ovviamente, una volta consegnati, uno dopo l'altro hanno iniziato a sgretolarsi; di fronte a delle buone intenzioni c'erano di contro delle cattive azioni da parte di chi, continuamente e sistematicamente, vuole speculare o seminare il seme del male in ogni azione, ancorché nobile. È di questi giorni addirittura la condanna del responsabile del procedimento. Anche quando la politica e le istituzioni sono all'altezza, poi ci si trova a doversi confrontare con il tessuto sociale ed imprenditoriale che purtroppo specula. Concludo, signora Presidente, facendo un'ultima considerazione che ho già fatto qualche anno fa. La brutta figura l'abbiamo fatta nella costruzione, ma la brutta figura all'Aquila l'abbiamo fatta anche quando, in primo grado, sono stati condannati degli scienziati perché non avevano previsto il terremoto: un terremoto non si può prevedere, quindi noi ribadiamo la nostra solidarietà a questi scienziati

al popolo dell'Aquila e degli altri Comuni del cratere. Vogliamo ricordare le 309 vittime, vogliamo ricordare le migliaia di feriti, vogliamo ricordare i ragazzi e le ragazze della Casa dello studente. Questa notte, alla fiaccolata, vi era uno striscione con una richiesta, un grido ancora

Noi non possiamo limitarci a ricordare e a fare l'ennesima commemorazione; dobbiamo continuare ad assumerci impegni, con la Commissione d'inchiesta,

È vero che in Cassazione vi è stata una certa sentenza, ma noi sappiamo perfettamente che molte di quelle vittime sono state causate anche dalle

in cui la ricostruzione ha faticato ed è stata costellata costantemente da episodi di malaffare, da tentativi di speculazione. La ricostruzione ha faticato per l'assoluta incertezza sui finanziamenti. Vorrei ricordare in questa sede che una delle prime questioni che abbiamo affrontato appena eletti riguardato il tentativo disperato di dare certezza al flusso di risorse per la ricostruzione dell'Aquila. Vorrei ricordare

di notte ancora si vede quel buco nero: è il buco nero di chi non ha saputo - e forse neanche voluto - per tempo essere vicino concretamente a quei cittadini e ricostruire il sesto centro storico d'Italia per monumentalità.

In questi anni, contraddistinti dai ritardi, vorrei ricordare che, anche oggi che i cantieri sono riaperti, mancano ancora molte risorse per completare la ricostruzione e restano molti nodi aperti. La disoccupazione all'Aquila è molto più alta della media italiana. Nonostante questi cantieri, noi continuiamo ad avere problemi molto seri. Vi è un problema enorme di identità. sede vogliamo rendere omaggio ai tanti cittadini che negli ultimi anni hanno continuato a sperare e anche a lottare per ricostruire la propria città e ridare un senso all'essere dell'Aquila e un'identità alla propria esistenza. Torno a ripetere che noi oggi esprimiamo solidarietà e ricordo, tuttavia quest'Assemblea dovrebbe assumersi, ancora una volta, degli impegni concreti perché la ricostruzione

Presidente, ci uniamo anche noi con commozione al ricordo di questo evento calamitoso di sette anni fa, che non ha lasciato scampo a molti abruzzesi, colpiti improvvisamente nel cuore della notte. Oltre alle vittime, dobbiamo ricordare tutte quelle persone e famiglie costrette ad allontanarsi dalla propria abitazione, perdendo tutto quello che fino a quel momento avevano costruito con i sacrifici di una vita. Il terremoto ha devastato il territorio abruzzese, a cominciare dall'Aquila, coinvolgendo anche circa 50 Comuni, alcuni dei quali sono stati completamente distrutti e, insieme a loro, anche buona parte dell'importante dell'importante patrimonio storico, artistico e architettonico di queste città. In ogni tragedia è comunque giusto rendere omaggio e riconoscere storie di grande professionalità, sacrificio, umanità e solidarietà. In questa sede vorrei ricordare tutte le Forze dell'ordine che hanno contribuito a fornire una prima assistenza alle popolazioni colpite sia in quei giorni, che nelle settimane immediatamente successive al 6 aprile 2009. Ricordo, inoltre, gli importanti aiuti che in Abruzzo arrivavano costantemente da parte delle ONLUS e del mondo del volontariato da tutta Italia, sotto forma sia di beni materiali di prima necessità, che di coinvolgimento in prima persona nelle operazioni di soccorso e assistenza. In particolare, vorrei ricordare il Corpo di polizia municipale di Roma che, nei mesi successivi al sisma, collaborò fattivamente con i Vigili urbani dell'Aquila e fornì attestazioni di sostegno e concreta e fattiva solidarietà al dramma abruzzese. Come ogni anno, anche la scorsa notte si è svolta la fiaccolata in ricordo delle 309 vittime del terremoto dell'Aquila. La manifestazione, promossa dai familiari delle vittime, è sempre un'occasione per chiedere verità e giustizia su questi fatti, nonostante il processo alla Commissione nazionale grandi rischi abbia avuto l'epilogo in Corte Il 20 novembre scorso è stata confermata la sentenza che ha assolto sei dei sette componenti che in primo grado erano stati condannati a sei anni di carcere per aver falsamente rassicurato gli aquilani e aver sottovalutato il rischio sismico al termine della riunione del 31 marzo 2009. L'unico a essere condannato a due anni è stato l'ex vice capo della Protezione civile. Vorrei concludere con un pensiero di speranza per il futuro. Nonostante le moltissime difficoltà incontrate nella ricostruzione dei territori colpiti, alcune importanti iniziative sono testimonianza di uno spirito e una voglia di ritornare alla normalità di una vita che si è improvvisamente spezzata sette anni fa.

il dolore per le tante vite cadute sotto le macerie del sisma. Da quel giorno sono passati sette anni di incalcolabile dolore e rabbia. Nessuna giustizia per le vittime innocenti e per i sopravvissuti. La paura difende e, invece, troppe persone nella mia città stavano dormendo e, forse, sognando o aspettando che quel pensiero che impediva il sonno sparisse dalla mente. Colleghi, non è facile mettersi nei panni di chi lo ha vissuto, eppure è possibile provare ad immaginare per capire ciò che è stato, sentire la lunghezza degli attimi, gli strilli di mura contorte, lo sbriciolarsi di un intonaco, il peso di una parete che ti ostruisce il passaggio, il dolore di un corpo lacerato, l'odore di polvere e calcinacci. È possibile provare a vivere un brutto sogno di questo tipo, ma con la consapevolezza di avere l'enorme privilegio negato agli aquilani di poterlo allontanare e tornare alla vita di sempre con i propri cari e all'interno della propria casa. Giusto e doveroso è il momento di ricordo in quest'Assemblea delle vittime innocenti del terremoto che flagellò in una notte il capoluogo dell'Abruzzo, ma per moltissime famiglie le «macerie» sono ancora lì, immobili come le lapidi del ricordo. Ringrazio i colleghi che hanno sottolineato in questa Assemblea la difficoltà economica che vive la popolazione, la difficoltà che vivono i tanti giovani disoccupati e le famiglie che devono pagare ingenti bollette e ancora continuano a pagare mutui per case distrutte. Nomi legati a volti e storie sono stati scanditi nel silenzio di questa notte, dopo il percorso di una fiaccolata che da sette anni è diventata l'appuntamento per tutti gli aquilani che, al suono interminabile dei 309 rintocchi, vivono un intreccio di emozioni difficile da comprendere, si uniscono al lutto ed alcuni ricevono forza per sperare di potercela fare. Sperano di poter rivedere la città più bella e più sicura, perché la perdita dei propri cari non sia stata vana e per i tanti giovani pieni di speranze, che ci hanno lasciato prematuramente in quella notte. L'Aquila è una ferita è una ferita aperta del Paese e non potrà rimarginarsi finché non emergeranno tutte le verità e finché non verrà fatta giustizia di tutti i soprusi e le illegalità che continuano ad essere fonte di lucro per pochi e di grande sofferenza e scoraggiamento per molti, ai quali fa male passeggiare tra quei mozziconi di edifici disperati, tra le infinite impalcature coperte di ruggine, alla ricerca di quei privilegiati palazzi che, tra nuvole di polvere fina, irrespirabile e maleodorante, lentamente rivedono l'antico splendore. Gli aquilani del cratere sismico sono stanchi di parole, di visibilità estemporanee, delle tante promesse non mantenute, dei fiumi di soldi malamente utilizzati per la ricostruzione e spero venga avviata al più presto la Commissione parlamentare

Per il 7° anniversario del terremoto dell'Aquila non basta che Guido Bertolaso, che ha voluto creare l'aspettativa all'Aquila dei massimi esperti italiani per rassicurare, continui a confermare ai microfoni di SkyTG24 la sua intenzione di rinunciare alla prescrizione nel processo Grandi

partendo dalla rivisitazioni di alcuni istituti giuridici, come la prescrizione e l'omicidio colposo, come ha giustamente affermato ieri Antonietta Centofanti. questo giorno deve diventare un grande momento nazionale di riflessione su sicurezza, trasparenza, partecipazione, corretta informazione e soprattutto onestà e legalità. Solo così sarà vera commemorazione.

Ricorre infatti il 7° anniversario del violento terremoto che ha colpito il capoluogo di Regione, con le sue 309 vittime e la devastazione di un intero territorio e del suo tessuto economico e sociale. Tante giovani vite sono state portate via, con il loro limpido corollario di speranze e di sogni, gettando nello sconforto più profondo intere famiglie e comunità. un dolore che ha attraversato inesorabile tutti questi anni e che si rinnova ogni 6 aprile con maggiore forza e intensità, un dolore profondo e incancellabile, un solco vivo nella nostra coscienza collettiva di uomini e donne. È difficile trovare le ragioni e la forza per andare avanti e per costruire, giorno dopo giorno, i presupposti necessari a riconnettersi con la vita quotidiana e i suoi riti. La ringrazio, quindi, Presidente, per aver fermato i lavori dell'Assemblea con un sentito minuto di cordoglio

Signora Presidente, senatrici e senatori, sette sono i vizi capitali, sette sono le virtù, sette sono state le piaghe d'Egitto, sette sono i colori dell'arcobaleno. Un'alternanza di gioie e di dolori sembra essere legata a questo numero. Sette sono ormai gli anni trascorsi da quella notte orrenda, che mai nessuno di noi riuscirà a dimenticare. Sono ancora molto vividi i ricordi e le emozioni, il boato, l'urlo dell'orco, la terra che trema, mia figlia che piange disperata e mi chiede che cosa sta accadendo, i giocattoli che le cadono addosso, la fuga da casa, la ricerca frenetica di notizie di parenti e amici. Poi la corsa verso Onna la terra di mio padre - da dove cominciavano a trapelare le prime notizie di morte e disperazione, con cui abbiamo imparato, per giorni, a fare i conti. Sembra assurdo, sembrava impossibile e invece è accaduto ed è tutto vero. Sette anni sembrano un tempo sufficiente per dimenticare, per andare avanti, ma non si può dimenticare. In molti di noi quel ricordo, il ricordo delle 309 vite spezzate, è ancora vivo. A tenerlo acceso contribuiscono sette anni di bugie, di mistificazioni, di speculazioni. Abbiamo dovuto fare i conti con le bugie del miracolo della ricostruzione del Governo Berlusconi, con l'efficientismo di facciata di Bertolaso, con le risate delle ore 3,32 e con le speculazioni legate alla ricostruzione. Abbiamo dovuto resistere alla deportazione in massa di 40.000 persone sulla costa,

Abbiamo dovuto fare i conti con la sentenza della Commissione grande rischi, altro schiaffo alla memoria delle nostre vittime, ai loro familiari e a una città ancora ferita, che viene ora sbeffeggiata dalle promesse di Bertolaso ai romani di compiere lo stesso miracolo dell'Aquila. Rinunci piuttosto alla prescrizione e consenta di verificare ogni responsabilità. Se siamo riusciti a sopravvivere a tutto questo, è grazie alla forza e alla tenacia che abbiamo saputo tirar fuori, per vedere la nostra città e i tanti comuni ricostruiti. Abbiamo lottato ogni giorno e i risultati si cominciano a vedere. In periferia la maggior parte degli aquilani è rientrata nelle abitazioni di sempre e il centro storico sta lentamente trovando una sua nuova grande bellezza. A ricostruzione ultimata avremo una delle città più belle d'Europa. Lo dobbiamo alla nostra gente, lo dobbiamo all'Italia, lo dobbiamo ai nostri giovani, a quelli che non ci sono più, che hanno perso la vita quel tragico 6 aprile e a chi c'è, perché è voluto tornare. Lo dobbiamo ai nostri figli, affinché possano ereditare una città accogliente e sicura e ai tanti giovani che continuano a volerla bella. Con questo spirito abbiamo questa notte portato le fiaccole del dolore e della speranza. Abbiamo partecipato in tanti alla fiaccolata per ricordare le 309 vittime innocenti, fino alle 3,32 a scandire i nomi: ogni nome, un rintocco della campana. C'è stato con noi anche il Governo con il sottosegretario alla Presidenza del consiglio De Vincenti, segno di vicinanza e affetto, e con il prefetto Tronca, che in quei giorni, di capo dei Vigili del fuoco, ci è stato vicino. Tanti erano i volontari, anche questa notte, anche questa mattina ad accompagnare il dolore con le fiaccole. Non chiedeteci di dimenticare quella notte, non chiedeteci di non raccontarla. Quella notte, i giorni che l'hanno preceduta, tutto quanto accaduto in questi sette anni, non è solo la nostra storia, ma un pezzo importante di storia d'Italia. In molti

tempo. A ricostruzione ultimata avremo una delle città più belle d'Europa. E le oltre 100 gru del centro storico sono un segno di speranza nel giorno del lutto. Noi

14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione

velocemente calendarizzata la mozione di sfiducia nei confronti del Governo. Signora Presidente, come lei può ricordare o come ricordo a me stesso, è prassi, quando un Capogruppo richiede la convocazione della Conferenza, che la stessa sia riunita. Non è accaduto nella giornata di ieri. Abbiamo atteso fino a questo momento che qualche cenno arrivasse dalla Presidenza, ma non è ancora avvenuto. Ieri abbiamo assistito alla comunicazione del ministro Gentiloni

Temo che si stiano banalizzando cose estremamente serie. La nostra richiesta di convocazione della Capigruppo è finalizzata alla messa in discussione della mozione di sfiducia al Governo e questo non può essere derubricato come un argomento di secondo livello:

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge del Governo sulle banche, che ci accingiamo a convertire, contiene alcune norme come quelle sulle cartolarizzazioni che, data la situazione a cui siamo pervenuti, potranno un po' aiutare senza comunque risolvere la questione gravissima dei crediti deteriorati che pesano sui bilanci del sistema bancario italiano e mettono piombo nelle ali all'attività creditizia. E tuttavia, dico Vi è un'altra norma assai più importante e incisiva, che è la riforma del credito cooperativo. Anche in questo caso mi viene da dire che lo schema funziona. C'è tuttavia, anche per effetto del lavoro svolto dalla Camera dei deputati, dei deputati, un passaggio che complica inutilmente le cose e credo vada lumeggiato. Questo passaggio è costituito dalla cosiddetta *way out* facilitata per le banche di credito cooperativo con capitale superiore ai 200 milioni e per altre che a queste, nel giro di sessanta giorni, si possono aggregare, attraverso il conferimento dell'azienda bancaria a una SpA, ovvero la vendita della medesima attività bancaria a una banca già esistente. Perché dico che questa norma non funziona? Non funziona perché non obbedisce alla logica che ha ispirato l'azione di Governo fin qui - e che abbiamo già ritrovato nella riforma delle banche popolari la quale tende ad accrescere la dimensione delle banche in modo tale da consentire economie di scala e maggiori efficienze gestionali a favore del loro consolidamento e della loro capacità di fare credito all'economia. In questo caso, qualora la *way out* venisse imboccata, noi avremmo una proliferazione di banche di dimensione microbica e, quindi, contraria all'impostazione generale. Tuttavia, siccome la norma è fatta male, è molto probabile che siano pochissime le banche di credito cooperativo che imboccheranno questa strada,

Questa misura - a mio parere - è impropria, perché costituisce *de facto* un'imposta senza dichiararsi tale: si parla di versamento, non d'imposta. Se avessimo voluto parlare d'imposta, avremmo dovuto definirla come imposta sostitutiva per affrancare le riserve indivisibili. Ma siccome non vogliamo affrancare le riserve indivisibili che restano in capo alla cooperativa, costringiamo ogni caso a fare questo versamento, che - a mio parere - è poco legittimo, perché costituisce una discriminazione a danno delle imprese cooperative che vogliano effettuare un'operazione di scorporo di ramo d'azienda, che viene fatto normalmente dalle società di capitali. Questa norma sbagliata ha, l'effetto positivo di scoraggiare le BCC dall'imboccare la via di uscita. Capite che siamo nel regno della tortuosità. Perché le scoraggia? L'intera riforma del credito cooperativo, positiva, si basa su un'analisi dei fatti inoppugnabile, e cioè le banche di credito cooperativo hanno un patrimonio netto mediamente rilevante, meglio di quello delle banche SpA - la media vuol dire che alcune non ce l'hanno - ma, rispetto ad esse, hanno anche una quantità di crediti deteriorati, e tra questi di sofferenze, più elevata e meno coperta dai fondi di svalutazione. Pertanto, nel sistema del credito cooperativo c'è un equilibrio tra il maggiore patrimonio e i minori fondi. si mette un balzello del 20 per cento del patrimonio su chi vuole cedere l'attività bancaria a una SpA, indebolisce pesantemente il patrimonio medesimo; restano i fondi di svalutazione insufficienti e un patrimonio indebolito.

Bisogna guardare i bilanci, e allora si scoprirebbe - per esempio - che la BCC di Cambiano - il cui consulente Nicola Rossi ha rivendicato, sul «Corriere della sera», la paternità della norma che ci viene oggi proposta scenderebbe da un patrimonio leggermente inferiore a quello medio delle BCC attuali

viene considerata debole, meritevole di soccorso, di ricapitalizzazione. E non solo: anche la copertura dei crediti deteriorati risulta largamente inferiore alle soglie indicate dalla vigilanza.

Naturalmente la norma è una opzione, non un obbligo, e quindi saranno i soci di queste cooperative a ragionare sulla convenienza o no di imboccare questa strada. Infatti, credo che all'atto del conferimento dell'attività bancaria nella SpA o della vendita a un'altra banca si apriranno due problemi, il primo dei quali sulla natura della cooperativa che resta.

spiegò che le banche di credito cooperativo non sono cooperative qualsiasi, ma sono imprese bancarie cooperative e cioè, nel momento in cui non hanno più attività creditizia nel proprio

Ma non è questo il punto principale, siamo realisti. Il punto principale è che, se dal 15 per cento delle attività ponderate per il rischio si vede il patrimonio calare sotto il 12 per cento, quando la quota

la domanda è la seguente: secondo voi, questo aumento di capitale sarà facile da collocare sul mercato in un momento in cui gli sportelli bancari vengono regalati, nel momento in cui quando si offrono 20 o 30 sportelli bancari si crea un problema a chi li deve acquistare? Chi sta facendo queste norme sa in che mondo vive o insegue delle ubbie e dei pensieri vaghi?

Stiamo parlando di banche - ripeto - e non di unioni civili o di letteratura. Se noi arriviamo a dover fare un aumento di capitale che sarà di difficile collocazione, dovremmo anche stabilire un valore

al mondo della finanza ben più collaudata nel tempo, con una reputazione più importante, si trattano in borsa al 50 per cento del valore patrimoniale.

una volta trasformata in SpA e pagate le imposte come si deve e non più come cooperativa, avrebbe un utile di meno di 4 milioni all'anno e, quindi, potrebbe valere una quarantina di milioni. cerca di collocare le azioni sul mercato, si deve anche fare uno sconto. Ricordo che il valore del patrimonio netto attuale di questa BCC è di 278 milioni

Detto questo, credo che voterò comunque a favore del provvedimento in esame, perché - come ho appena finito di illustrare - si tratta di una cosa sbagliata, ma così sbagliata che non verrà utilizzata per cui rimarrà in piedi

le dico subito che questa riforma non ci piace, ci lascia perplessi e ci preoccupa. Ci preoccupa perché le banche di credito cooperativo nascono per servire il territorio,

che si uniscono non ne fanno certo una capitalizzata. Dovranno arrivare comunque capitali dall'esterno e quelli che arriveranno guideranno *holding* e banche di credito cooperativo secondo principi estranei ai principi mutualistici di queste banche. Andavano riformate le banche di credito cooperativo? Certamente sì, perché magari sono troppo soggette ai condizionamenti della politica e dei politici, ma da questo punto di vista non è stato fatto nulla. Rimane tutto uguale. Soprattutto non è stato fatto nulla dal punto di vista della riforma degli organi di controllo: parlo naturalmente di Banca d'Italia e Consob. Consob. Signori, fin quando avremo una Banca d'Italia controllata dalle stesse banche che deve controllare, si ripeteranno continuamente i casi drammatici come quello della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca che hanno bruciato 16 miliardi di euro dei risparmiatori senza che gli organi di controllo muovessero un dito, ovviamente in termini di efficacia della loro azione di controllo. Di controllo. Di riforma della Banca d'Italia, invece, non si parla affatto. E questo non deve stupire, perché una riforma della Banca d'Italia che risolva il suo conflitto di interessi sarebbe nell'interesse dei cittadini, ma non nell'interesse del sistema bancario. E questo è un Governo che interviene solo con provvedimenti a favore del sistema bancario. I regali fatti dal Governo e dalla maggioranza alle più grandi banche del nostro Paese ormai non si contano più ve ne elenco alcuni (ma l'elenco sarebbe lunghissimo): siamo partiti dal decreto IMU-Bankitalia che ha regalato 7,5 miliardi alle banche principali del nostro Paese e ogni anno stacca un assegno in termini di dividendi dai 300 ai 400 milioni di euro che vengono percepiti indebitamente. Non sono mai stati percepiti nella storia della Repubblica italiana prima di questo decreto-legge. E non parliamo poi delle imposte ridotte sul *capital gain* contenute nel provvedimento. E i cittadini ringraziano. Poi c'è stata la cosiddetta *bad bank*, cioè la garanzia dello Stato sui crediti deteriorati. Ma perché non diciamo anche una parola sui dividendi di miliardi e miliardi che queste banche distribuiscono ai propri azionisti, prima di parlare di *bad bank*? E perché non parliamo di *bad bank* anche per i crediti deteriorati di altri settori importanti dell'economia? Pensiamo alle piccole e medie imprese. Quanti crediti deteriorati hanno le piccole e medie imprese su cui ci sarebbe eguale dignità di intervento? avete reintrodotto l'anatocismo. Ecco, di anatocismo in Italia se ne sentiva veramente la mancanza. C'era la gente che andava in piazza chiedendo al Governo di reintrodurre l'anatocismo. L'anatocismo era ed è vietato ai sensi dell'articolo 120 del testo unico bancario, almeno fino a questo provvedimento. Avete poi accorciato i tempi per il recupero delle perdite su sofferenze: era a diciotto anni, poi a cinque e poi a un anno solo. Avete fatto il decreto sulle banche popolari, che consente ora di poterle scalare e che ha gettato sul lastrico oltre 200.000 risparmiatori. Avete avuto Avete avuto il coraggio di proporre la perdita della prima casa per chi ovviamente ha stipulato un contratto di mutuo, dopo solo sette ritardi nel pagamento delle rate, senza passare dal giudice. Ovviamente i cittadini ringraziano per questi provvedimenti straordinari, fatti pensando proprio all'interesse del cittadino. Avete recepito, senza colpo ferire, il *bail in* e avete perfino prorogato, senza alcuna gara pubblica, la concessione dell'autostrada Padova-Brescia. E questo conferisce un vantaggio indebito di due miliardi di euro, che sono soldi pubblici che passano dalle casse dello Stato alle tasche dei privati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E allora andiamo a vedere chi sono questi privati: azionista di maggioranza della concessionaria Padova-Brescia è una banca. Guarda la coincidenza! Noi cosa proponiamo? Abbiamo avanzato le nostre proposte. innanzitutto di mantenere gli istituti bancari con le loro specifiche peculiarità. Vogliamo evitare un modello unico di SpA

che è un progetto, e quindi una volontà, che parte dallo stesso mondo delle banche di credito cooperativo. Ma allora, se così fosse, aderirebbero comunque. Che necessità c'è, dunque, di imporre l'obbligo? Abbiamo proposto anche una SpA capogruppo partecipata esclusivamente dalle banche di credito cooperativo, sostituendo la forma sociale SpA in un consorzio di banche di credito cooperativo, perché stranamente il Governo si è dimenticato di introdurre efficaci barriere all'ingresso di capitali estranei al mondo della cooperazione. In conclusione, signora il decreto-legge sulle banche di credito cooperativo è inutile per i cittadini, per i clienti, per i territori, ma soprattutto è inutile per gli oltre 1.230.000 soci di questi istituti. rischia di portare alla desertificazione del credito alla piccola impresa nel nostro Paese. Al contrario, è utilissimo ai grandi gruppi bancari, che vogliono mettere le mani sulla *holding* e soprattutto sulla raccolta delle banche di credito cooperativo. Concludo dunque con una domanda, che ho già rivolto in Commissione, senza ottenere una risposta. Siccome non trovo altra logica e siccome avete frapposto le fondazioni tra i finanziatori della politica e la politica, per rendere opachi questi rapporti, vi chiedo:

certamente non è facile intervenire in pochi minuti su un provvedimento così complesso, sul quale non c'è stata offerta alcuna opportunità di discussione e modifica. è già intervenuto ieri il senatore Carraro, e condivido perfettamente tutto ciò che ha detto e la denuncia che ha fatto in ordine all'assurdità del metodo utilizzato, che però nasconde naturalmente una utilità

Vorrei anche dire al senatore Mucchetti, che esprimeva delle perplessità in ordine alla possibilità di offrire sul mercato futuri aumenti di capitale, che già Palazzo Chigi sta provvedendo. Ieri vi è stata in quella sede

preoccupati dell'impossibilità di mandare sul mercato aumenti di capitale sensibili per alcuni importanti istituti bancari nazionali, stanno elaborando un nuovo intervento legislativo, l'ennesimo, che sarebbe il quarto a questo punto. E spero che questo quarto intervento venga quantomeno assegnato, come si suol dire in termini legislativi, al Senato perché possa essere qui discusso: almeno noi potremmo dire qualcosa in merito. Questo sta a denunciare come l'intervento complessivo e globale del Governo sul sistema bancario sia dovuto sempre a motivazioni episodiche ed emotive e non a un quadro complessivo e coordinato. Dissi a suo tempo che era la seconda grande occasione sprecata da questo Governo, a paragone con un più famoso Governo precedente: la prima fu quella di non aver affidato a un

la riforma del sistema bancario italiano. Tutto ciò ha introdotto solamente elementi parziali, sui quali ci si potrebbe anche divertire a scoprire alcune amenità, alcune perle, come si dice in gergo.

nel senso complessivo e generale del Paese. Questi sono provvedimenti che servono non all'economia del Paese, ma solamente a un settore, e sono fatti nella omissione di una considerazione: le banche non sono l'economia del Paese,

nel 1996-1997 con la vicenda del Banco di Napoli. La cartolarizzazione è l'estrapolazione dei crediti di dubbio esito e il posizionamento in una banca che io chiamo «banca dei cattivi» (per non usare quei termini inglesi che non mi sono molto congeniali).

debitori delle banche, delle piccole imprese, e non solamente a vantaggio di coloro che andranno ad acquisire questi pacchetti e a specularci sopra (e nei prossimi mesi sapremo chi sono). Faccio una piccola notazione su una perla di questo provvedimento. L'articolo 4, al comma 1, lettera *a),* dice che «i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile». una cosa assolutamente ovvia! Chi comprerebbe mai un dubbio esito a un valore superiore al valore contabile? Bisognava mettere un paletto al contrario: bisognava dire "che ha un valore non inferiore a una

l'ufficiale giudiziario dietro la porta di casa senza sapere per quanto è stato ceduto il suo credito e quanto gli viene richiesto per la finale definizione del debito.

debiti ceduti e sottoposti alle procedure agevolate di cui alle disposizioni in esame, anche perché non è stato posto neanche un paletto temporale alle indicazioni delle sofferenze di dubbi esiti. Oggi come oggi, le banche possono inserire nella cosiddetta banca dei cattivi (ossia tra i crediti crediti da cedere) qualsiasi loro credito e debito di terzi, perché rientra nella loro assoluta discrezionalità comporre questi pacchetti, come avvenne - ripeto - nel 1996 con il caso del Banco di Napoli. Quindi, ci apprestiamo ad assistere a un fenomeno speculativo incredibile di banche che compongono i pacchetti da cedere e di società che li comprano con la garanzia dello Stato

amenità, buone per il mercato bancario e finanziario europeo, ma non certo per la struttura socio‑economica del nostro Paese). Saranno quindi inseriti in questi pacchetti e ceduti; si troveranno un creditore diverso dalla banca da cui avevano preso il denaro, con cui non

nell'ambito del mercato immobiliare nazionale, un gravissimo *vulnus* alle ordinarie transazioni. È infatti chiaro che, avendo solamente un onere fisso di 200 euro per poter pagare la tassa di acquisto di un immobile, chi è normalmente sul mercato si asterrà dal farlo, attendendo l'opportunità

su cui dovremmo contare per avere una ripresa economica e non certo sui vantaggi che arrechiamo al settore bancario, penalizzando invece l'economia reale. Si tratta di un problema di impostazione filosofica

e interessi singoli. Una cosa sono le *lobby*, che possono anche essere normate per legge, un'altra sono gli interessi singoli che sono alla base di tutti i provvedimenti, dai

c'è stato un dibattito molto ampio in Aula, che segue quello altrettanto ampio avvenuto in Commissione. Nonostante il poco tempo a disposizione e nonostante il fatto che il Senato sia stato parzialmente escluso

stato significativo. Stiamo per aggiungere un altro mattone alla costruzione di un grande edificio e c'è coscienza di ciò tra i colleghi. Senza interloquire, la prima cosa che mi sento di contestare al senatore D'Alì è che manchi un quadro complessivo e coordinato e che si tratti della somma di tanti episodi. Cercherò nel corso del mio intervento di dimostrare il contrario, avendo una visione d'insieme strategica che penso faccia la differenza in questi temi. temi. La costruzione di questo grande edificio ha come oggetto proprio la riforma del sistema bancario perché il dibattito in questa sede si è molto concentrato sul tema delle banche di credito cooperativo, che era il tema più ghiotto, ma non ci dimentichiamo che parliamo anche di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze tema rilevante e significativo che ha visto un confronto importante in Europa e anche su questo voglio tornare - del regime fiscale relativo alle procedure di crisi e della gestione collettiva del risparmio. Questa è la dimensione dei provvedimenti che affrontiamo quando ragioniamo di riforma del sistema bancario. Il nostro *Premier* qualche giorno fa ci ricordava che il 2016 è l'anno in cui l'Italia deve sistemare definitivamente la propria questione bancaria, che non è grave come in altri Paesi, ma ha dei profili di problematicità. Stiamo lavorando da qualche settimana pancia a terra tutti i santi giorni per avere una soluzione che sia compatibile con le regole, che dia tranquillità e garanzie a investitori e risparmiatori e certezza agli istituti di credito. verso i quali sta tendendo il Governo e anche noi, come Parlamento, cerchiamo di dare, per quanto possibile, un contributo a tutto questo. Quando parliamo di riforma del sistema bancario non possiamo prescindere dal fatto che qui non si tratta di una questione solo italiana, italiana, ma europea e il tema di fondo è quello dell'unione bancaria europea. Sappiamo che tutto nasce dalla crisi del 2007, dalla crisi del 2007, che ha palesato la necessità di armonizzare in tutta l'Unione europea, ma soprattutto nella zona euro, la regolamentazione delle attività bancarie e la vigilanza delle stesse, perché perché si è formata la convinzione che un'errata valutazione dei rischi da parte del settore bancario stesso avrebbe potuto compromettere la stabilità finanziaria degli Stati membri. Quindi si arriva al giugno del 2012, quando si ha un cambio di prospettiva netto e il Consiglio europeo decide di spezzare il circolo vizioso che esiste tra le banche e il debito sovrano. Per fare questo, si utilizza lo strumento dell'Unione bancaria, che si regge fondamentalmente su tre pilastri. Il primo è il meccanismo unico di vigilanza, che decolla subito; il secondo è il meccanismo di risoluzione unico, che è diventato operativo dal primo gennaio 2016, e il terzo è quello del fondo di risoluzione unico, che invece, nelle prospettive che ci vengono delineate, dovrà entrare in vigore nel 2023. 2023. Il senso del lavoro che stiamo cercando di fare, che vuole avere una visione organica, è quello di affrontare anche il terzo tema in fase ascendente, proprio perché ci rendiamo conto che è strettamente collegato agli altri due e ha delle ripercussioni significative,

in termini reali, al ruolo che sono chiamati a svolgere i Parlamenti nazionali nel percorso di costruzione della legislazione europea.

Mi permetto quindi di ricordare quanto sostenuto l'anno scorso in riferimento al decreto-legge n. perché, nel ripercorrere il quadro complessivo, non possiamo perdere di vista lo sfondo che caratterizza l'azione del Governo e anche il contributo offerto dal Parlamento. Enumerando le misure adottate in materia creditizia dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, oggi come allora sono convinto che le azioni indirizzate alle banche e agli intermediari finanziari costituiscano uno strumento fondamentale di politica economica,

alle banche. Questa è una lettura assolutamente riduttiva e quanto mai fuorviante: si tratta invece di intervenire su un settore nevralgico dell'economia, tanto più in una congiuntura di ripresa, ovvero in un momento in cui le risorse aggiuntive fornite dal credito sono assolutamente strategiche per il futuro. Un anno fa ritenevo che nel contesto completamente mutato dell'Unione bancaria, dei tassi negativi,

aumentando l'erogazione del credito. Non è mai simpatico citarsi, ma devo dire che proprio allora addossavamo alle banche italiane una grandissima responsabilità. «tocca adesso a tutti i banchieri italiani meritare lo sforzo e la prontezza del legislatore, per sostenere, con innovazione e fantasia, rischio imprenditoriale e sfida del futuro, la ripresa dell'economia». Sostenevo questo perché denunciavamo e sottolineavamo come, in controtendenza rispetto a quanto sarebbe stato auspicabile, alcune banche italiane avessero utilizzato le risorse a bassissimo costo del per restituire alla BCE le linee di finanziamento precedentemente assorbite ad un costo superiore a quelle dei LTRO. Si passava da 0,25 a 0,05 ma il rapporto era sempre di 1 a 5. E noi evidenziavamo quei limiti del sistema dicendo che, adesso che avevamo creato le condizioni perché questo non capitasse più, e quindi richiamando alle proprie responsabilità le banche, volevano che vi fosse un contributo a quella ripresa che noi troviamo assolutamente fondamentale per il lavoro che stiamo svolgendo. Allo stesso tempo, davo atto al Governo di aver superato le colonne d'Ercole di un bacino ristretto autoreferenziale, quale quello del settore bancario, con la riforma delle banche popolari. a tale innovazione si aggiunge oggi il nuovo assetto della galassia del credito cooperativo. Personalmente sono soddisfatto del testo accolto dalla Camera dei deputati, poiché l'impianto del progetto della Federcasse è stato confermato. Sono garantite alternative all'adesione al gruppo delle BCC, ma senza stravolgere i principi della cooperazione. Perché dico che sono contento? Permettetemi di ricordare con un po' di orgoglio che il progetto di riforma è stato seguito dalla Commissione finanze sin sin dall'inizio. È stato oggetto di un seminario svoltosi qui in Senato con l'omologa Commissione della Camera e presenta dei contenuti di interesse generale. Oltre tutto, furono proprio le banche di credito cooperativo che (all'interno dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario che permise di avere una fotografia positiva di quello che era, ed è, il sistema bancario in Italia), memori di quanto era successo, da un lato alle banche popolari, più volte sollecitate ad autoriformarsi

una via per trovare un protocollo d'intesa significativo, avevano innescato un processo di autoriforma e avevano deciso di discutere questo processo con il Parlamento. Gli elementi fondamentali emersi in quel seminario si ritrovano assolutamente tutti nel decreto legge presentato alla nostra attenzione. Il credito cooperativo rappresenta un elemento di peculiarità e si è parlato, soprattutto nel dibattito in Commissione, di una biodiversità finanziaria, che ha bisogno di essere sostenuta in un momento di rapidi mutamenti. Non lo si fa con le risorse pubbliche, ma attraverso una impalcatura giuridica che risponde all'esigenza di vigilanza sistemica e salvaguarda le singole realtà economiche vicine al territorio, mette a fattore comune servizi ed esperienze ed è una risposta forte del sistema della politica. Si cambia la prospettiva ma è certamente una risposta all'altezza dei tempi che viviamo. Ed è la risposta migliore ad alcune delle critiche che sentivo in questa sede. Ma voglio utilizzare non le mie parole, bensì quanto detto ieri da Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative,

La famosa *way out* che viene concessa alle BCC che non vogliono aderire al gruppo unico sarà quella di lasciare le riserve indivisibili nella casa madre, e conferire l'attività bancaria in una Spa dietro pagamento di una imposta». «questo salva i principi, e offre la possibilità a chi non vuole stare nel gruppo unico di trovare una nuova soluzione; ma penso che saranno molto poche le BCC che non aderiranno al gruppo unico, perché i tempi sono difficili e richiedono un gruppo unico che faccia da ombrello e dia protezione». Egli esprime con ciò un giudizio assolutamente positivo del lavoro che è stato fatto. Dal dibattito sulle banche popolari e sul credito cooperativo emergono certamente delle voci preoccupate sul destino delle aziende italiane, sull'ingresso degli investitori stranieri o comunque estranei alle logiche naturali e agli interessi economici italiani. In una condizione statica di eredità soddisfacente, tale insistenza non sarebbe stata giustificata. Al contrario, dopo la recessione, tutto il sistema bancario e finanziario si è riorientato e si sta riorganizzando a regole variate ma con bilanci pesanti e aumenti di capitale privato che, complessivamente, ammontano a circa 50 miliardi. Lo snodo di questi anni si presenta quindi veramente cruciale. Il Governo ha ritenuto importante superare vincoli giuridici grazie ai quali una certa tipologia di attività creditizia aveva preso forma e si era sviluppata. In futuro non sarà così: spetta adesso al banchiere tornare a fare il proprio mestiere, sapendo che gli attori del mercato sono più forti, che la vigilanza sistemica è in campo e che la tutela del risparmio non arriva più a coprire con le finanze pubbliche la totalità dei soggetti investitori ma solo i depositari. Le novità normative del decreto in esame si inseriscono in una congiuntura che segna quindi un miglioramento dell'attività bancaria grazie al superamento della condizione tecnica della lunga recessione e grazie alla conferma,

Nel 2015, infatti, si sono manifestati segnali di ripresa in Italia e per le banche l'andamento dei nuovi prestiti è stato particolarmente vivace nel comparto dei mutui, dove si è registrato il sostanziale raddoppio di flussi complessivamente erogati alle famiglie (con poco più del 30 per cento di operazioni di surroga), ed è stato promettente anche nel comparto delle imprese, dove i nuovi impieghi sono cresciuti dell'11,6 per cento su base annua. Grazie al perdurare di queste dinamiche nel corso di buona parte dell'anno passato, verso la fine del 2015 anche lo *stock* complessivo di prestiti in essere all'economia (compresa la pubblica amministrazione) ha smesso di contrarsi e ha registrato valori lievemente positivi: questi sono dati di fatto. Noi tutti sappiamo però che il peso relativo sistemico dei crediti deteriorati e degli accantonamenti fatti dalle banche mettono in forse la capacità di irrobustire la crescita economica, come denunciato anche nel *country report* sull'Italia, fatto dall'Unione europea. È alla luce di simili considerazioni che dobbiamo tornare con la mente a tutte le misure poste in essere, perché solo così possiamo renderci conto del tipo di azione che si sta svolgendo con quest'ultimo mattone (come l'avevo definito la cessione delle quote di Banca d'Italia, la riforma delle banche popolari, le norme sui requisiti patrimoniali, l'impalcatura della vigilanza europea, l'autoriforma del sistema delle banche di credito cooperativo, il regime di deducibilità di perdite su crediti, le misure di accelerazione del recupero dei crediti e, per ultimo, i programmi di finanziamento della BCE e gli interventi di acquisto di titoli pubblici, anche detenuti da banche, della stessa autorità di Francoforte.

sugli strumenti in campo. I membri della Commissione, che hanno seguito tutta la questione attraverso un'indagine conoscitiva, hanno osservato il percorso con particolare attenzione. Di recente è stato autorevolmente sostenuto che tale confronto poteva essere condotto con maggiore decisione; al contempo è chiaro a tutti che il peso relativo dello *stock* e del flusso dei crediti deteriorati sulle banche non può essere affrontato con strumenti ordinari e di lungo periodo. Al dicembre 2015 i crediti in sofferenza rilevanti, cioè quelli non rettificati dalle banche ammontano non a 202 miliardi ma a 84 miliardi,

Il decreto interviene quindi in una prospettiva di politica economica: la liquidità messa a disposizione dalla BCE non si trasforma in nuovo credito; i bilanci delle banche sono fortemente appesantiti dalle perdite e dai crediti deteriorati; le misure di stabilità sistemica richiedono accantonamenti sui crediti robusti con capitale di qualità e collaterale costoso. Da qui l'esigenza indifferibile e urgente di attivare il mercato dei titoli cartolarizzati con sottostanti crediti bancari. Su questo aspetto la novità della Camera di estendere anche agli intermediari finanziari la facoltà di cartolarizzare crediti assistiti dalla garanzia dello Stato appare rilevante nella prospettiva di irrobustire il mercato dei titoli cartolarizzati. Non vi è dubbio, quindi, che la garanzia dello Stato, nei limiti del decreto-legge (limiti derivanti dalla trattativa con l'Unione europea), sembra operare con effettività e incisività (forse non quella auspicata ma è comunque significativa), ed è uno strumento aggiuntivo al mercato. Penso che alcuni elementi nuovi dei mesi scorsi richiedano comunque una riflessione un po' più ampia. Gli investitori hanno velocemente abbandonato le posizioni sulle banche quotate immaginando nuove debolezze strutturali e fragilità sistemiche, che non apparivano giustificate, soprattutto alla luce della fotografia che avevamo fatto sul sistema bancario italiano. A un livello totalmente diverso, e cioè quello dei clienti e dei risparmiatori italiani, si è diffusa la stessa sfiducia nelle banche e nelle istituzioni finanziarie, dopo la crisi delle quattro banche - e l'applicazione parziale del meccanismo di salvataggio interno anche a causa di un'informazione giornalistica troppo spesso superficiale se non terroristica. Permettetemi di dire, con voce chiara, che le cose non sono come vengono dipinte: noi abbiamo un sistema bancario italiano sano con alcune criticità e stiamo seguendo con attenzione particolare, soprattutto nell'interlocuzione che c'è con l'Unione europea, tutte le questioni che si riverberano direttamente e che non accettiamo passivamente come calate dall'alto.

attenzione alla fase ascendente per cercare di seguire i processi e non subirli con logiche di recriminazione che non servono a nulla.

allora a riaffermare il concetto espresso dal noto scrittore indo-britannico, riformulandolo e attualizzandolo alla luce delle considerazioni che facevo all'inizio del mio intervento, conscio dei miei limiti e senza voler assolutamente pormi in competizione con lui, concludendo che solo un'idea di Europa fondata su diritti certi per tutti permetterà il superamento di un concetto di Europa basato su doveri solo per alcuni, perché nel difficile equilibrio tra diritti e doveri auspichiamo che tutti gli Stati siano uguali e non ci sia nessuno più uguale degli altri. *(Applausi

sul merito del provvedimento, che però non colgono l'elemento essenziale di una serie di interventi che rafforzano l'intero sistema bancario; interventi come questo delle BCC che riprende le linee guida elaborate dal mondo delle banche di credito cooperativo e che si muove all'interno delle due coordinate fondamentali: il rafforzamento del sistema, da una parte superando la parcellizzazione, la frammentazione e quindi la debolezza strutturale; dall'altra, mantenendo le finalità di credito cooperativo. Quindi ribadisco

oggi compiamo un altro passo importante su un tema come quello del sistema bancario che - ricordo - è l'unico canale che alimenta la nostra economia, il nostro sistema di imprese. Segniamo imprese. Segniamo un ulteriore passo in avanti per poter affrontare al meglio le questioni che abbiamo ancora davanti, e cioè la partita dei crediti deteriorati, che però oggi può essere vista e affrontata in un quadro sicuramente più stabile e più forte, tenuto anche conto dell'attuale difficoltà di reperimento di capitale in un quadro di mercato molto difficile. Da questo punto di vista, la patrimonializzazione patrimonializzazione e l'impiego di risorse private e non pubbliche per rafforzare il sistema è un altro elemento a favore. Per questo giudico molto positivamente il provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

e cioè sulla scelta di procedere in questa materia per decreto-legge. Naturalmente è stata una scelta opinabile è ovvio - e non è stupefacente che sia stata una scelta sottoposta a numerose valutazioni critiche anche nel corso di questa discussione. semplicemente provare a dire che non si è trattato, tuttavia, di una scelta priva di motivazioni che hanno qualche fondamento razionale. Chissà perché bisogna per forza rovinare i tentativi di discutere seriamente. Dev'essere una malattia.

norme fiscali sui contributi ricevuti a titolo di liberalità da soggetti in procedura concorsuale) e che costituiscono

troppo lungo) di preparazione sia in sede nazionale (riforma delle banche di credito cooperativo) sia in sede europea (le altre due scelte fondamentali). Cosicché, appena definite le intese su ognuno di questi punti, sia con i soggetti che chiameremo di natura economico-sociale sia con i soggetti istituzionali (soprattutto gli organismi comunitari), si è scelto di adottare le soluzioni definite per decreto-legge al fine di accelerare il processo di entrata in vigore di questo complesso di norme di particolare rilievo. Era infatti divenuto urgente un intervento di rafforzamento del sistema delle banche di credito cooperativo anche per favorire il consolidamento patrimoniale delle banche stesse e, in particolare, di quelle in difficoltà. Ho ascoltato un intervento in cui

A mio giudizio il numero delle banche di credito cooperativo che hanno serie difficoltà è inferiore ma in ogni caso vi è una forte esigenza di consolidamento e di rafforzamento cui la soluzione contenuta nel decreto cerca di dare una risposta. Così come era diventata urgente, dopo quasi un anno di confronto e di trattativa in sede europea, la soluzione di apporre una garanzia di Stato sulle cartolarizzazioni che abbiano come sottostante sofferenze bancarie e crediti deteriorati,

Appena definita la soluzione europea, abbiamo scelto di agire per decreto-legge, perché bisogna far partire immediatamente il processo che consentirà ad una quota, a mio giudizio significativa, di queste sofferenze di essere collocate sul mercato a condizioni più appetibili. Bisogna infatti sapere, torno ad insistere su questo argomento, che è una ragione di particolare debolezza. Il nostro sistema bancario ha i profili e le caratteristiche che qui sono stati richiamati. Non è vero che si tratti del sistema bancario più debole in Europa, ma è tendenzialmente vero il contrario. Non abbiamo dovuto mettere soldi dei contribuenti per rafforzare il sistema. Queste sono tutte affermazioni infondate. Siamo però un Paese nel quale abbiamo conosciuto una recessione molto lunga nel tempo, tale per cui abbiamo perso, tra il 2008 e il 2014, il 2014, 9 punti di prodotto interno lordo e 10 punti di reddito medio *procapite*. È del tutto evidente che le imprese che lavorano per il mercato interno hanno dovuto fare i conti con un mercato che si è venuto drammaticamente restringendo.

Mauro Maria Marino). È chiaro allora che se vogliamo fare in modo che l'orientamento di politica monetaria ultraespansiva della Banca centrale europea si trasmetta all'economia reale, producendo più investimenti più posti di lavoro, dobbiamo cercare di affrontare il tema delle sofferenze. Il tema delle sofferenze bancarie si affronta attraverso molte iniziative, ma una di queste è la costruzione, anche in Italia, di un mercato delle sofferenze bancarie che non c'è. La garanzia di Stato può fornire per un segmento di questo mercato l'impulso a nascere e a costituirsi. Per fare che cosa? Per risolvere i problemi delle banche perché astrattamente siamo

Per uscire dal *credit crunch* bisogna ridurre le sofferenze in maniera tale che le banche abbiano le risorse necessarie per tornare a fare il loro mestiere, cioè tornare a fare credito alle imprese, perché senza credito non si ha

decreto era ottenere dal Senato il consenso necessario per confermare il testo uscito dalla Camera, non soltanto perché fare il contrario e rendere necessaria una terza lettura metterebbe a rischio la conversione definitiva di questo decreto (e non ce ne è davvero bisogno), quanto e soprattutto perché soprattutto perché consideriamo che le soluzioni adottate alla Camera risolvano positivamente le due questioni fondamentali che in senso critico si sono proposte sul testo originario del decreto.

per le banche di credito cooperativo che non intendano aderire ad un gruppo bancario nazionale cooperativo e una debolezza nel riconoscimento delle peculiarità territoriali, dell'esperienza e della natura delle banche di credito cooperativo. Questi erano i due difetti fondamentali del testo del decreto-legge. Prima di arrivare, e concludere rapidamente, a questi due punti fatemi fare un'osservazione di carattere generale. Certamente sulla via d'uscita c'è stata una grande discussione e il Parlamento è intervenuto modificando radicalmente il testo originario del decreto, ma è un errore a mio giudizio concentrare così ossessivamente l'attenzione sulla via d'uscita, facendo perdere il senso - scusate cioè della soluzione rappresentata dalla costituzione del grande gruppo bancario o dei grandi gruppi bancari cooperativi. Questa è la soluzione attraverso la quale le singole banche di credito cooperativo confermano la loro natura di banche ispirate al principio di mutualità, confermano la loro natura di banche particolarmente radicate su specifiche porzioni di territorio, ma si collegano e si aggregano nazionalmente per affrontare problemi, a partire dalle dotazioni patrimoniali di capitale, che sono affrontabili in una in una chiave di maggiore aggregazione. Ora, io parlo di gruppi bancari cooperativi nazionali, non necessariamente di gruppo, perché chi conosce la consistenza del patrimonio netto del movimento delle banche di credito cooperativo sa che il limite che abbiamo fissato non necessariamente descrive l'obbligo di fatto, per legge, di costituire un gruppo unico; altra cosa è avere un orientamento tendenzialmente favorevole ad un'aggregazione la più ampia possibile. Confermo che l'orientamento del Governo, coerente in questo senso con quello di Federcasse e del movimento delle banche di credito cooperativo, è a favore della più ampia aggregazione, con l'obiettivo di un'unica aggregazione,

senza dire per forza che chi non condivide la nostra opinione è caratterizzato da insipienza e non sa cosa sta facendo, forse faremmo un passo nella direzione giusta. Io non dico che chi ha avanzato critiche non sa cosa dice; sa cosa dice ed avanza critiche che meritano di essere discusse.

con l'orizzonte nelle opzioni politiche (ma non nel vincolo di legge) che se ne costituisca anche uno solo, possiamo noi vietare e togliere una via d'uscita o condizionarla esclusivamente alla totale devoluzione delle riserve delle banche di credito cooperativo attraverso ciò che è reso necessario dalla legge sulla cooperazione (non sulle banche di credito cooperativo)? La cooperativa che si scioglie è allora pensato che la soluzione del gruppo unico per legge, cioè imposto dal vincolo della legge, fosse una soluzione non percorribile. Per questa ragione abbiamo teso a tenere molto alte le soglie, in particolare la soglia del miliardo, in un contesto nel quale è stato necessario trovare una via d'uscita. Riconosco che la via d'uscita che il Governo aveva individuato nel testo originario era una soluzione sbagliata; l'abbiamo riconosciuto apertamente. Forse andrebbe considerato questo elemento, perché non era tanto sbagliata con specifico riferimento alle banche di credito cooperativo, ma era una soluzione che metteva in discussione un principio fondamentale del movimento cooperativo nel suo complesso: la cooperativa la puoi sciogliere, se vuoi, e la puoi trasformare in SpA, ma, ma, per piacere, le riserve che in parte significativa sono frutto delle agevolazioni fiscali che lo Stato riconosce sacrosantamente, in applicazione della Costituzione, alle cooperative le devolvi al fondo mutualistico. Il rischio che questo precedente delle banche di credito cooperativo, che aveva una sua giustificazione, attraesse tutto il movimento della cooperazione ci ha indotti a considerare altre soluzioni. La soluzione che abbiamo presentato a questo proposito, discussa alla Camera e approvata, è a nostro avviso soddisfacente, perché non elimina l'affrancamento delle riserve. La cooperativa rimane cooperativa ed è titolare delle sue riserve fintantoché non deciderà di sciogliersi; a quel punto, le riserve saranno devolute al fondo mutualistico. non intende aderire al gruppo cooperativo grande e ha le dimensioni previste dalla norma (200 milioni di euro di patrimonio netto) questa cooperativa può scegliere, rimanendo cooperativa (poi vedremo quello che

(perché bisogna costituire il grande gruppo di credito cooperativo e non possiamo dare molto tempo per questa decisione). Questa soluzione prevede il mantenimento di un versamento - come è stato chiamato nel testo - del 20 per cento non delle riserve o del capitale (come è stato detto), ma del ma del patrimonio netto. Perché abbiamo mantenuto questa norma? È una scelta opinabile, naturalmente, ma è una scelta che, da un lato,

nel momento in cui fa un trasferimento di ramo d'azienda in una SpA qualcosa deve restituire di quel vantaggio. Ecco perché è un versamento e non una generica imposta. Naturalmente sul numero si poteva discutere (20 o

eventualmente ognuna di esse trascinandone qualcuna delle altre. Prevedo, come hanno detto in molti, che saranno poche, ma questa via d'uscita era assolutamente necessaria per fare in modo che, da un lato, ci fosse tutto l'intervento pubblico, tutta la regolazione favorevole a un orientamento di aggregazione al massimo livello, senza negare, dall'altro, che, sia pure pagando un prezzo importante, fosse possibile percorrere una qualche soluzione alternativa. Da questo punto di vista, a mio giudizio, la soluzione che abbiamo trovato, quindi, ha una sua logica. E ha una sua logica - lo voglio dire al senatore Molinari - anche

seconda criticità. Nella norma originaria non c'era un sufficiente riconoscimento delle peculiarità territoriali del movimento delle banche di credito cooperativo. Non c'era questo riconoscimento per quella componente del movimento delle banche di credito cooperativo che ha le più straordinarie peculiarità: Bolzano e, per certi aspetti non identici, Trento.

di utilizzare quello che prevede questa norma, allora dovranno fare un'operazione di scorporo di quelle banche di credito cooperativo che non operano nella Provincia di Trento, altrimenti dovranno fare altre scelte: potranno fare un sottogruppo o altre cose, ma non certamente usare la norma così com'è, che fa esplicito riferimento alle banche che hanno sede e operano nella Provincia in questione. Per Bolzano è così, per Trento oggi non è così. Naturalmente c'era però il problema di andare oltre. Bolzano e Trento hanno peculiarità, che però sono presenti, sia pure in modo non così marcato, anche in altre realtà. Qui abbiamo adottato una soluzione che, secondo me, si fa male a sottovalutare. Abbiamo stabilito che le banche di credito cooperativo di una certa entità territoriale che lo ritengano, possono costituire un sottogruppo in forma di

con assoluta tranquillità, si è orientato a difendere in Senato un testo che, a nostro avviso, il Parlamento ha modificato in modo radicale su punti che erano critici e che oggi lo sono, se non altro, un po' di meno.

onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2298, di conversione del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori per la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge di riforma delle banche di credito cooperativo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Per consentire l'inizio della chiama alle ore 17, si è stabilito che la seduta odierna sarà unica. La discussione sulla fiducia, per la quale è stata ripartita un'ora e dieci minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi, avrà inizio alle ore 14. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. Al termine del voto di fiducia è convocata la Conferenza dei Capigruppo. Sospendo

finestra"). Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 5 aprile 2016 Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Federica GUIDI dalla carica di Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di reggere ad interim il predetto Dicastero. F. *to* Matteo Renzi». Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà. Signora Presidente, parlando di fiducia su un provvedimento, non c'è dubbio che ci dobbiamo chiedere se questo Governo meriti ancora fiducia oppure no. A noi, colleghi di quest'Aula, sembra quasi sembra quasi ridicolo dover parlare di fiducia su un provvedimento parziale e settoriale, quando sappiamo che ci sono due mozioni di sfiducia sul Governo in generale e che, se passassero quelle, non avrebbe più senso parlare di fiducia su un provvedimento. Dovendo parlare però del provvedimento, dovremmo anche chiederci dove ci sta portando questo Governo.

fintanto che qualche membro del Governo non fosse disposto ad ascoltare. Ma, proprio per quello che dirò,

Il guaio è che tutto il Paese sta vivendo questo disagio e questa scollatura, con un Governo che sembrava aver dato fiducia e voler provare strade nuove.

di Galli della Loggia inizia proprio con queste parole: «C'era un Renzi che ci piaceva». Potremmo anche non leggere tutto il resto, perché «c'era»

Nel testo, che è abbastanza puntuale, dell'editoriale del «Corriere della

«Era di sinistra» significa che portava avanti tematiche, prospettive e soluzioni che la sinistra

alla parola chiave che definisce la sinistra nella storia, è «partecipazione». Tra il centralismo, l'uomo solo al comando e il sistema democratico partecipativo la sinistra ha sempre piantato paletti: sinistra vuol dire allargare la platea delle decisioni, renderle più accettabili, creare

ma non si può prescindere da una partecipazione istituzionale. Nella riforma istituzionale Renzi ha cancellato sostanzialmente il potere legislativo delle Regioni: non esiste più la potestà legislativa

chiaro che c'è una difesa molto più strenua da parte delle Province autonome e delle Regioni a Statuto speciale. Ma, tornando al Parlamento, il Parlamento non conta più nulla.

non darà più fiducie, non darà più indirizzi politici, non voterà più il bilancio dello Stato. Un Parlamento eletto non viene più chiamato ad esprimersi per mano di un Governo il cui Presidente del Consiglio non è nemmeno un eletto. Qui si possono aprire scenari per giuristi amanti della narrativa politica di questo Paese: è possibile che un Governo non eletto metta in scacco e - a questo punto - fuorigioco un Parlamento eletto (nel bene o nel male, con una buona legge o con una cattiva legge)? Perché dico questo? Perché nella fiducia nella fiducia i numeri sono importanti e quando un Governo arriva e dice: «Pongo la fiducia», ciò significa: «Non mi interessa conoscere la vostra opinione. Non mi interessa la vostra partecipazione al confezionamento della normativa e del provvedimento che si sta discutendo. Prendete oppure lasciate». In un momento storico che lascia ambiti oscuri

il centrodestra mai è stato così sfilacciato, porre la questione di fiducia sa solo di ricatto: poiché non sarete in grado di fare altro e digovernare senza di me,

disegni di legge di iniziativa parlamentare sono pressoché ininfluenti. Il Governo ha l'arroganza di adottare un decreto

il tanto bistrattato Monti, che ne chiese di fiducie, non pose mai la fiducia su disegni di legge di iniziativa governativa. Stiamo assistendo a un'*escalation* spaventosa di concentrazione di poteri.

del lavoro che la sinistra ha provato ad ostacolare, sulla riforma della pubblica amministrazione e anche sulla legge di stabilità del 2015, della quale mi pare che qualche marachella sia emersa in questi giorni, a proposito di parenti o non

in mano soltanto ad un partito, che esprimerà un Governo monocolore, che poi esprimerà, a cascata, tutte le alte cariche di controllo e di governo, tra cui il Presidente della Repubblica, abbiamo capito in che *cul de sac* ci siamo infilati.

Si capisce benissimo che questo è un anno elettorale per cui si pensa a qualche manovrina, ma non possiamo andare avanti a furbate e, soprattutto, non possiamo lasciare in mano ad un Governo

coniato un*modus operandi* che poi è stato scalfito, come qualche scrittore ha riportato bene. Puoi anche fare il furbo, ma le cose non durano in eterno; puoi ingannare poca gente per tanto tempo oppure puoi ingannare tanta gente per poco tempo,

dovute calendarizzare anche le mozioni di sfiducia presentate da alcuni Gruppi politici.

non era possibile programmare un voto di sfiducia nei prossimi giorni fino all'esito del voto di fiducia che si avrà oggi sul provvedimento che, come ho detto, noi

o nel girone dilettantistico, come ha sempre cercato di fare da vent'anni e più a questa parte, quando ha contribuito

non può essere esaminato, perché il Governo non può chiedere 200 fiducie. Semmai, dopo questo voto di fiducia, i Gruppi che lo ritenessero necessario dovranno ripresentare perché non è possibile promuovere fiducie o sfiducie preventive. Il Parlamento oggi si esprimerà e deciderà se questo Governo debba andare a casa oppure se è legittimato perché oggi andremo a votare

nostro Gruppo ritiene che la riforma costituzionale sia necessaria, che il bicameralismo ormai debba essere superato e che ci voglia un'unica un'unica Camera che, ovviamente, abbia la possibilità di legiferare in maniera istantanea, pronta, adatta ai tempi e per essere competitivi con l'Europa

che c'è un Presidente del Consiglio non legittimato. La Costituzione lo legittima: una volta avuto l'incarico dal Presidente delle Repubblica e la fiducia dai due rami del Parlamento si è il Presidente del Consiglio,

della nostra Costituzione, i magistrati sono soggetti soltanto alla legge e alle leggi che il Parlamento fa e sapere e vedere che dei semplici funzionari pubblici,

tribuna. Solo in Italia un giudice audisce o ascolta un Ministro, non succede da nessun'altra parte del mondo. D'altronde, signora Presidente, in Italia abbiamo avuto anche Presidenti della Repubblica che non erano parlamentari

è un tema che sta particolarmente a cuore ai cittadini, alle imprese ed ai nostri tessuti sociali ed economici. Lo è soprattutto adesso, nella grande fase di trasformazione che stiamo attraversando, in cui c'è grande attenzione affinché quello italiano sia un sistema stabile, in grado, cioè, di garantire pienamente i correntisti e gli investitori e di stimolare e supportare in maniera intelligente il mondo delle imprese. Provengo da una terra dove il credito cooperativo da sempre costituisce uno strumento prezioso al servizio della popolazione, dell'economia, del territorio e della sua crescita. Tuttavia, questo decreto-legge, quantomeno nella sua versione originaria, rischiava di farne perdere questa funzione. Per questo voglio ringraziare il Governo che ha saputo tenere in giusta considerazione le nostre sollecitazioni, con l'intento di tutelare un sistema che ha una sua specificità ma che soprattutto funziona, svolgendo un prezioso compito anche di carattere sociale. È importante procedere con le riforme, con la modernizzazione del sistema Italia, ma nel farlo bisogna sempre avere grande cura per evitare che quello che funziona possa essere smantellato, mantenendo sistemi e strutture consolidate e vincenti. Non posso, allora, che salutare con grande favore le parole che il vice ministro Morando ha speso questa mattina in quest'Aula nella sua replica, parlando di Bolzano e di Trento, sottolineando, da un lato, come nella norma originaria mancasse il sufficiente riconoscimento delle specificità del movimento delle banche di credito cooperativo di Bolzano; dall'altro, il fatto che le Raiffeisen sono sì chiamate a contribuire agli obiettivi di carattere generale, ma attraverso un percorso autonomo e di piena tutela della loro particolarità. Il sistema cooperativo del nostro territorio affonda le sue radici nella storia ed è ormai presente da più di È un modello più simile a quello anglosassone che alla tradizione, altrettanto importante, del credito cooperativo italiano. In 107 dei 116 Comuni della Provincia di Bolzano troviamo gli sportelli della Raiffeisen a servizio del cittadino, con 47 banche, 62.000 associati e con una quota di mercato del 48

e che ha permesso al nostro sistema economico e sociale, a cominciare dall'ambito agricolo, di crescere, di svilupparsi e di superare tanti momenti di difficoltà. In generale, il nostro territorio è storicamente legato e anche caratterizzato dal principio della cooperazione che ha rappresentato una base e un pilastro per la gestione di situazioni di crisi nell'ultimo secolo. La piena adesione ai valori e ai principi mutualistici rappresentato la bussola che ha sempre guidato le scelte del movimento del credito cooperativo sudtirolese e in questo vi sono anche similitudini con quello di Trento, così come il Vice Ministro ha giustamente sottolineato. Durante la discussione generale, il senatore Panizza ha ben illustrato le caratteristiche del nostro sistema, i suoi numeri e il modo in cui interagisce con l'intero tessuto economico e sociale. Mi preme tuttavia economico e sociale. Mi preme tuttavia rimarcare ancora due elementi: il primo è la straordinaria funzione di supporto che ha svolto soprattutto negli anni più duri della crisi economica, perché senza il credito cooperativo molte aziende, forse, non ci sarebbero più. Il secondo è che, con il suo radicamento, finanche nelle più piccole realtà di montagna, il credito cooperativo svolge una funzione di presidio territoriale, garantendo servizi fondamentali per prevenire lo spopolamento e l'impoverimento dei territori. Pensiamo solamente alla funzione di supplenza che in futuro sarà chiamata a compiere a fronte della chiusura di diversi uffici postali. Insomma, se non fossero state recepite molte delle nostre sollecitazioni, si sarebbe generata una spirale negativa che avrebbe interessato anche il tessuto sociale. Credo che questa storia e i valori che la animano non possano essere cancellati, ma meritino invece di essere rilanciati.

e dalla trattazione molto rapida che abbiamo potuto riservargli che la sua storia fosse già scritta, come del resto ha confermato, durante i brevi lavori, lo stesso vice ministro Morando. Mi limito adesso ad alcune rapidissime considerazioni sul contenuto, sui tre temi principali che secondo me caratterizzano questo provvedimento. Per quanto riguarda le BCC, anche apprezzando il fatto che almeno questa volta, contrariamente a quanto era accaduto con la riforma delle banche popolari, i diretti interessati siano stati coinvolti ed abbiano potuto almeno esprimere e vedere in parte accolta la propria idea di autoriforma, ritengo che questo sia un ulteriore passo verso la standardizzazione dell'ecosistema bancario.

Questo renderà tutto il sistema del credito, a mio avviso, meno resistente e meno in grado di rispondere a possibili futuri *shock* sistemici. Ho anche apprezzato l'intervento di ieri del senatore Collina, nella prima fase della discussione, nel quale il senatore ci ha fatto una bella lettura sulle nuove regole europee e sul *bail in* che però, se può avere qualche attinenza con la seconda questione che tratta questo provvedimento, secondo me con la riforma delle BCC ha poco a che fare. Se nello stesso discorso

un mercato drogato, con delle cartolarizzazioni che speriamo non finiscano mai per vie traverse in mano a chi non è in grado di capire ciò che sta comprando. Ma i recenti fatti direbbero di essere un po' più prudenti su questo argomento.

L'ultima questione è quella dell'anatocismo. Dico che a tal riguardo avete avuto davvero la possibilità di chiudere la questione in maniera pulita e a favore dei cittadini e - a mio avviso - è stata sprecata, con una soluzione che magari migliora il caos assoluto di fronte al quale ci siamo

e giunge da noi in Senato per una sostanziale ratifica priva di qualsiasi possibilità di intervento correttivo, perché il Governo ritiene suo pieno diritto difendere una scelta di cui è convinto anche con l'apposizione della fiducia.

Intanto per due anni abbiamo portato avanti un'indagine conoscitiva sul sistema bancario, nel corso della quale sono stati discussi tutti gli aspetti critici del sistema stesso: dall'eccessiva quantità di crediti deteriorati, affrontata in parte in questo provvedimento, fino alla possibilità di adozione di una Glass-Steagall Act italiana,

sul sistema di garanzia dei depositi, sull'unione bancaria, sulla vigilanza unica: insomma su tutti quei temi che riguardano il mondo bancario. il livello di approfondimento raggiunto possa esserci riconosciuto senza grossi problemi, e lo dico da persona dell'opposizione che riconosce i meriti in generale del lavoro

una seconda volta, la considero un incidente spiacevole. Ma la terza volta esprime la volontà chiara di escludere il ramo del Parlamento che maggiormente ha approfondito i temi bancari dal poter dare il proprio contributo al miglioramento dei provvedimenti che vertono temi. Forse chi ha esaminato un argomento con un certo livello di approfondimento è meglio che taccia, per non disturbare i manovratori. Che cos'è questo? È il superamento del bicameralismo? Il collega che mi ha preceduto ha parlato della riforma costituzionale: tutto molto interessante, ma attualmente il sistema è ancora bicamerale e soprattutto, se qualcuno svolge un'attività così approfondita su un determinato tema, magari avrebbe diritto di poter dire la sua, e non solo per ascoltare la propria voce, ma anche per poter vedere recepite alcune sollecitazioni che giustamente vengono dal mondo esterno dal mondo esterno che vive tali problematiche e, nel caso specifico, dal mondo esterno del credito. Io ritengo che questo svilisca l'attività di tutti i parlamentari di questo ramo del Parlamento, e non solo di quelli dell'opposizione. Mi auguro onestamente che il comportamento del Governo non esprima invece un giudizio sul livello di affidabilità nei confronti di chi lavora nelle Commissioni di merito, perché in questo caso, visto che di ciò parliamo, non posso che dire che la sfiducia sarebbe reciproca. Presidente, colleghi, ci troviamo dinanzi all'ennesimo provvedimento del Governo sul fronte bancario in poco più di un anno. una situazione che mi fa pensare alla celeberrima locuzione latina *gutta cavat lapidem:* proprio come la goccia che imperterrita agisce su uno stesso punto della roccia, questo Governo ha dimostrato un certo iperattivismo sul tema bancario, caratterizzato da vari interventi mirati a modificarne il sistema a proprio uso e consumo. Naturalmente Palazzo Chigi si ostina a parlare di riforme, ma in realtà definirei questi provvedimenti una vera scalata al potere del sistema bancario, a danno dei risparmiatori; insomma un tentativo di pluralizzare la celeberrima frase «abbiamo una banca» in «abbiamo molte banche». Ma si sa che i proprietari della nuova ditta pensano più in grande dei vecchi gestori. Da Fassino a Renzi il PD prosegue con il controllo della finanza italiana. Avete iniziato con il decreto-legge sulla *governance* delle banche popolari, trasformando in società per azioni quelle che avevano un attivo superiore agli 8 miliardi. E avete proseguito con l'ormai tristemente noto decreto salva banche, che ha ridotto in rovina ben 10.500 obbligazionisti, truffati per una somma di 340 milioni di euro, a cui è stato promesso un risarcimento di soli 100 milioni, meno di un terzo del valore della truffa, e i cui termini sono scaduti già da una settimana senza che abbiate fatto nulla. Si tratta di provvedimenti che non posso chiamare riforme, per la discutibile natura e la fumosa motivazione; provvedimenti, quindi, i cui benefici sono ancora tutti da verificare, a differenza, però, degli effetti negativi, che invece permangono e si protraggono con conseguenze sull'intero Paese. Infatti, proprio due giorni fa, l'ISTAT ha dichiarato un rialzo della pressione fiscale dello 0,2 per cento, a causa del precedente citato decreto-legge salva banche. Proprio un grande risultato! I Governi della sinistra che si sono susseguiti sono stati capaci di aumentare le tasse agli italiani dal 42,5 per cento dell'ultimo Esecutivo del presidente Berlusconi per cento dell'amministratore unico Renzi. Sono certo che gli italiani sappiano ben leggere questi dati. Prova ne è che, dagli ultimi sondaggi, il centrodestra è maggioranza relativa nel Paese e ha superato la sinistra di potere. Mi chiedo, quindi, se la maggioranza sia davvero convinta di accordare, ancora una volta, la fiducia su un provvedimento della stessa natura e riguardo un settore che impiega 135 miliardi

Già solo la mera elencazione di questi dati può dare un'idea di come le banche di credito cooperativo ricoprano un ruolo basilare per l'economia e siano una realtà fortemente e storicamente legata al territorio. Proprio da questi soggetti deriva poco più del 22 per cento dei prestiti erogati ad artigiani e piccole imprese italiane. E in Italia, dove le piccole e medie imprese sono la forza e la spina dorsale dell'economia nazionale, avere banche che conoscono davvero il territorio e gli imprenditori è un fattore decisivo di sviluppo e crescita del nostro Paese. Di fatti, sono state le banche di prossimità (le popolari e le cooperative, appunto), lontane dalla speculazione internazionale e dai *trading* aggressivi, a permettere al sistema finanziario italiano di resistere durante gli anni più difficili della nostra crisi. Sono assolutamente convinto che il sistema delle banche cooperative necessitasse di miglioramenti per garantirne la sopravvivenza nel mercato finanziario di oggi, ma non sono certo i modi e i tempi voluti dal Governo che permettono tutto ciò. Non si spiega, infatti, l'urgenza che ha richiesto l'uso del decreto-legge, considerando che le banche di con un indice di patrimonializzazione più elevato della media, e solo una ventina di esse sono considerabili a rischio. Non si spiega, infatti, la creazione del gruppo bancario cooperativo, di credito cooperativo di cui si definisce, quale unico requisito, il patrimonio netto di un miliardo e nulla, invece, si dice sui poteri e sui compiti di questo soggetto, la cui definizione è rinviata allo statuto. Non si spiega, infatti, la soglia per il cosiddetto *way out* posta a 200 milioni di euro, un limite fissato senza alcuna giustificazione, che ricorda molto la soglia di 8 miliardi prevista nel provvedimento sulle banche popolari. È una clausola incomprensibile e per nulla attrattiva,

Infine, mi chiedo cosa c'entri con la riforma delle banche di credito cooperativo la confusione creata con l'anomalo contenuto dell'articolo 17 del provvedimento, con il quale si interviene su una pluralità disomogenea di temi. in tema di anatocismo, assegnando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi, proseguendo con il regresso per il mancato pagamento di un assegno bancario e - per concludere - fornendo l'interpretazione alle norme sui pagamenti diversi da quelli in contanti. di una vera confusione, ma si sa che essa è la prassi con cui agisce questo Governo: è la sua migliore alleata e lo strumento che gli permette di perseguire i propri interessi. Concludo ricordando a quest'Assemblea che l'articolo 45 della nostra Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, ma - soprattutto - prescrive che «La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità Ebbene, il provvedimento in esame non rispetta alcuna delle caratteristiche espressamente previste dalla nostra Costituzione, ma il rapporto problematico tra l'Esecutivo e la nostra Carta e la questione di fiducia è diventata lo strumento con cui se ne fa beffa.

ci apprestiamo a convertire ha recepito gran parte delle proposte che, dopo mesi di lavoro, il credito cooperativo ha messo a punto e che, ancora prima della scorsa estate, aveva consegnato alle autorità competenti - Governo e Banca d'Italia con l'ambizione di disegnare un nuovo modello di integrazione a rete non mutuato da altre realtà omologhe europee. Infatti, altrove, in Europa, quei modelli organizzativi si erano perfezionati nell'arco di anni, forse decenni, e sulle riforme di quei modelli organizzativi, come ad esempio il Crédit Agricole o le Raiffeisen, già citati, nessun Governo si sarebbe mai sognato di ricorrere alla decretazione d'urgenza e - peggio ancora - di porre la questione di fiducia.

Va però ricordato che proprio nel gennaio 2015 il Governo, varando il famoso decreto sulla sbagliatissima riforma delle banche popolari, provò a inserire anche il provvedimento sulle Quel decreto-legge, se fosse stato convertito nella versione originaria, avrebbe cambiato radicalmente il volto alla cooperazione mutualistica di credito e posto le premesse per un inarrestabile declino del loro ruolo sul territorio. Ecco il punto vero: il loro ruolo sul territorio, vicino alle economie, quelle reali, e alle famiglie che in questi anni hanno visto perdere la loro capacità economica, che si è tradotta spesso poi in sofferenza bancaria. tornerò poi sul tema delle sofferenze bancarie perché rischia di passare in secondo piano, nel dibattito economico e anche politico, una questione che invece segnerà pesantemente la vita sociale delle persone, delle famiglie e delle imprese nei prossimi anni. Come dicevo, nonostante questo, le banche del territorio sono riuscite a contenere e a fare da argine a quella drammatica crisi. Lo ha ricordato stamattina il vice ministro Morando: 10 punti di PIL persi in pochi anni, bruciati da una finanza, che non è la finanza delle BCC o delle banche cooperative. Giova ricordare che le banche più piccole hanno 17 miliardi di quelle sofferenze, quelle medie ne hanno 39 e le prime 5 ne hanno 133. Questi sono i numeri veri, i miliardi di sofferenze a fronte di un credito erogato dalle banche piccole e medie che si attesta intorno ai 170 miliardi di euro: 170 miliardi sono i soldi che danno e 17 miliardi sono le sofferenze. Questa era la grande anomalia italiana che si voleva correggere. Nel correggerla però altri l'hanno corretta meglio di noi - rischiamo di mandare in fumo un intero sistema che ha accompagnato l'unica vera grande crescita del nostro Paese che è avvenuta dal dopoguerra fino a pochi anni fa. Si conferma che tra la mutualità prevalente e la mutualità non prevalente si gioca ancora lo straordinario ruolo delle cooperative, della cooperazione al fianco delle piccole imprese, insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale. Si conferma il drammatico errore fatto dal Governo con il decreto dello scorso anno che fissava - lo ha ricordato bene il collega Galimberti prima - la soglia dimensionale di 8 miliardi di attivo per il mantenimento dello *status* di banca cooperativa, che tradotto voleva dire: chi proprio non può fare a meno di utilizzare lo strumento della solidarietà e della cooperazione, si deve fermare a 8 miliardi di attivi, perché il mercato è fatto solo per chi della solidarietà e della cooperazione può anche non interessarsi. A questo riguardo ho accolto come un ravvedimento operoso la disponibilità del vice ministro Morando ad ascoltare le proposte contenute in emendamenti e ordini del giorno che abbiamo valutato in Commissione e auspico che rapidamente il Governo rimedi a un macroscopico errore, considerando anche il fatto che è riuscito a violare tutto il violabile possibile, dall'articolo

quantomeno, quella della vigilanza, che fissa a 30 miliardi di attivo il tetto entro il quale devono poter stare coerentemente le cooperative che fanno credito. Signora Presidente, noi Conservatori e Riformisti da tempo diciamo di essere preoccupati dalla tendenza che il Governo porta avanti, perché sono tutti interventi frettolosi: prima le banche popolari -

si è intervenuti malamente sulla questione dei crediti deteriorati, come ho detto all'inizio del mio intervento. Abbiamo sottovalutato i tempi e il modo del passaggio al *bail in* e ancora incombe su di noi questo tragico errore. C'è una maniera di procedere disarticolata e, quindi, pericolosa. La pericolosità emergerà quando le famiglie e le imprese faranno i conti con la gestione di queste sofferenze che, affidate ad altre società finanziarie che le comprano per pochissimo,

Persino il Ministro dell'economia e delle finanze oggi è costretto ad ammetterlo: nulla di ciò che avete fatto porta sollievo all'economia. E allora vi lambiccate intorno ai numeri della cooperazione bancaria,

per sostenere invece, convintamente, il coraggioso e virtuoso processo delle BCC, che vogliamo accompagnare verso un'economia che sappia riportare la persona al centro dell'attività economica, anche perché in quei territori, insieme alle BCC, alle imprese imprese e alle famiglie ci viviamo, ci lavoriamo e siamo qui a rappresentare.

Il Senato è ancora una volta escluso dall'attività emendativa. La sua prerogativa di incidere sull'*iter* legislativo è disattesa e resa vana. Il tempo c'era, ma ha prevalso la paura; la paura del Governo, che è consapevole di non aver più i numeri nel Paese e nel Parlamento, essendo Verdini dipendente, tiene unita una finta maggioranza in Senato, solo con il voto di fiducia e il timore di molti parlamentari di andare a casa, più rappresentativi dei cittadini, ma solo ed esclusivamente di se stessi. Pur non condividendo le scelte del Governo, abbiamo partecipato con nostre proposte emendative sia alla Camera dei deputati quindi, non ci siamo limitati ad un'azione puramente critica. In Commissione finanze e tesoro, il Governo ha accolto alcuni nostri ordini del giorno, ovviamente troppo poco per modificare tutte le nostre perplessità e contrarietà sull'intero provvedimento. La serietà e la competenza del vice ministro Morando non sono motivi sufficienti per far modificare la valutazione nettamente negativa della Lega Nord sull'azione di governo di questo Esecutivo.

i risparmi dei cittadini saranno più al sicuro? Le scelte del Governo tutelano o penalizzano i risparmiatori? Le imprese - soprattutto le piccole e gli artigiani - e le famiglie avranno più facile accesso al credito? Siamo convinti di no e aggiungo, purtroppo, che siamo convinti che non sarà così. Nessuno vuole il peggio: la situazione è troppo grave per poterlo fare. Siamo convinti che la fragilità del sistema bancario sia in parte dovuta alla cattiva gestione di chi sedeva e siede in alcuni consigli di amministrazione, ma in gran parte è colpa delle scelte della politica italiana.

al sistema dominante, quello tedesco. Così facendo, però, non lo state riformando, ma lo state uccidendo. In Europa non esiste un sistema di micro e piccole imprese come il nostro. Qual è stata la vostra risposta? Questo modello va modificato, è anacronistico. Così facendo, le microimprese, che hanno fatto la fortuna del nostro Paese, stanno morendo a migliaia. In Europa, poi, il sistema bancario si regge su pochi grandi gruppi. Qual è stata la vostra risposta? Il modello italiano è superato, diamo il via alle aggregazioni. Uccidiamo il sistema ricco, complesso e competitivo dell'Italia perché così ai piani alti europei dicono deve essere fatto. Ma chi, in questi anni di crisi profonda, ha fatto più credito al nostro sistema produttivo? Chi ha cercato di tenerlo in vita? Proprio le banche popolari e le banche di credito cooperativo. Lo riconoscete anche voi. Lo dice anche Banca d'Italia. Ma lo dite come se avessero commesso un errore. Hanno fatto troppo credito a famiglie e imprese. Questa è la vostra assurda accusa. accusa. Ma cos'altro dovrebbero fare le banche per sostenere lo sviluppo e l'occupazione? Vendere prodotti finanziari? Questo è il vostro modello di banca? La verità è che, con le vostre riforme delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, non abbiamo alcuna certezza che il sistema sarà più solido. Abbiamo la sola certezza che perderemo un modello tutto italiano, costruito in più di cento anni di storia. Oggi si sancisce in quest'Aula un colpo gravissimo al sistema mutualistico e cooperativo del credito italiano. Vi assumete una gravissima responsabilità. Il risultato finale sarà meno credito e più fallimenti, meno sviluppo, meno occupazione, e la perdita di contatto del credito con il territorio. Il modello «banche più grandi uguale banche più solide» è tutto da dimostrare. Monte dei Paschi insegna, e così la Banca Popolare di Vicenza. Molti risparmiatori sono disperati, nella totale indifferenza del Governo. Ci chiedono una Commissione d'inchiesta. La istituiremo? Quando? Cosa aspettiamo? La fine della legislatura? In questo provvedimento avete anche codificato per legge l'anatocismo. Avete stabilito quando si può applicare e quando non sia possibile farlo. Avete stabilito la dose minima di anatocismo applicabile dalle banche. Non credo fosse questa la scelta giusta da fare. L'avete codificato, e non cancellato. Questa riforma è anche viziata dal solito tentativo del vostro Governo di favorire qualcuno e di non fare le regole uguali per tutti. La norma del *way out* (o via di fuga) ne è l'ennesimo esempio. Avete preso una decisione, ma non l'avete portata fino in fondo. Volete creare una unica *holding* di tutte le banche di credito cooperativo perché ritenete saranno più competitive? Ma almeno non cedete alla solita tentazione di fare favori agli amici del "giglio magico" o del Presidente del Consiglio. Qual è il senso della norma del *way out* per le banche di credito cooperativo con patrimonio netto superiore ai 200 milioni? Non ce l'avete ancora spiegato, e forse per pudore. Ci avete spiegato tanti altri aspetti, ma non questo. Avete Avete fatto sorgere il legittimo dubbio che volevate favorire alcune banche. Quali? Quelle toscane, quella di Cambiano, quelle renziane? Papà Boschi, papà Lotti, Verdini: sono questi i banchieri di riferimento per le scelte del Governo? Siete sempre moralisti con i processi degli altri, mai con quelli che interessano la vostra parte politica; sempre a denunciare il conflitto d'interessi, ma in realtà vedete sempre e solo la pagliuzza nell'occhio degli altri e mai la trave nel vostro. un Governo pieno di figli di banchieri ed ex banchieri, che promuove provvedimenti *ad hoc* per favorire i propri sodali, ma sempre con la faccia tosta di indignarvi se qualcuno si permette di farvelo notare. Il caso Tempa Rossa insegna. Ma si sa, a voi tutto è permesso. Pensate piuttosto a risarcire i risparmiatori che hanno perso i soldi di una vita con il vostro decreto salva banche. Questa è una priorità che state disattendendo. Datavi una mossa, perché non solo non avete più la fiducia dei cittadini, ma state ormai provocando una rabbia sempre più diffusa. Sono ogni giorno di più coloro che non sono più disposti a farsi prendere in giro dalle chiacchiere del Presidente del Consiglio. Noi non abbiamo alcuna fiducia che queste scelte offriranno vantaggi alle famiglie e alle imprese italiane. Non abbiamo alcuna fiducia in questo Governo e soprattutto nel Presidente del Consiglio. Noi non vogliamo essere vostri complici. La Lega Nord voterà contro questo provvedimento e l'ennesima richiesta di fiducia da parte del Governo. MPL))*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe e cari colleghi, è davvero con rammarico che oggi affrontiamo ancora una volta la tematica relativa al settore bancario,

alla base qualunque ragionamento e qualsivoglia capacità o possibilità di mediazione parlamentare rispetto a un settore che, invece, è di assoluta importanza, anzi fondamentale per la vita del Paese, che angustia la gran parte dei cittadini italiani e assilla la maggior parte delle famiglie italiane. Anziché affrontare il tema in maniera ampia, scevra anche da condizionamenti che spesso ci derivano dall'appartenenza a un Gruppo di maggioranza o di minoranza, a una parte o all'altra dell'Emiciclo - è materia fondamentale, è carne viva nella società e nell'economia del nostro Paese

Quando il Governo si blinda con la fiducia non è un'azione di fiducia chiesta al Parlamento - al nostro Senato in questo caso - ma è chiaramente un'indicazione di sfiducia nei confronti dei propri stessi parlamentari. I parlamentari di maggioranza oggi sono chiamati a dare ancora una volta carta bianca rispetto a ciò che si è operato in parte nell'altro ramo del Parlamento e in parte - devo nelle stanze chiuse del Governo. Lo debbo dire, signora Presidente: in materia bancaria, ben quattro decreti-legge negli ultimi quattro mesi hanno tutto il sapore, il significato, la sgradevole sensazione che le decisioni assunte dal Governo non fossero esattamente la libera determinazione di una linea da condurre, né la libera determinazione di una scelta giusta o sbagliata, assunta sulla base di propri elementi e valutazioni, ma fossero sempre decisioni a rincorrere perlomeno stati di crisi urgenti. Le risposte

Buccarella).* Per tutelare il risparmiatore truffato si stanzia una somma a ristoro assolutamente insufficiente, ma non la si eroga neppure perché la matrigna Europa ce lo impedirebbe. Poi, guarda caso, interviene Margrethe Vestager, la nostra commissaria per la concorrenza, a dire che è assolutamente lecito lecito fare gli arbitrati a livello statuale, a livello di ogni singola Nazione, per poter ristorare i danni subiti. E, nonostante l'intervento della altre volte odiosa commissaria Vestager, noi non interveniamo. E allora questa Europa quando ci conviene è cattiva e quando non ci conviene non lo è. Questo è un Governo che interviene per decretazione di volta in volta, che interviene di volta in volta a chiedere la fiducia sui provvedimenti senza fare poi i decreti attuativi rispetto

è stato anche autolesionista nelle dichiarazioni che ha reso: si è assunto delle responsabilità che in verità, se avesse avuto un po' di coraggio, non si sarebbe neanche dovuto assumere. E dire che lui è bravo a fare lo scaricabarili e, ma in questo caso non lo ha fatto, pur di salvare - udite, udite udite - i forti. Forti con i deboli e deboli con i forti. Non si poteva toccare la Banca d'Italia, attenzione: quello è un tempio. un tempio. La Banca d'Italia, negli ultimi vent'anni, non ha fatto altro che cercare di salvare il sistema. Vogliamo vederlo un attimo? Scusate se faccio faccio entrare nell'Aula alta del Parlamento italiano problemi che riguardano la Banca d'Italia. Bene: in questi ultimi vent'anni, ogni volta che si manifestava una sacca di crisi, ogni volta che emergeva una banca, anzi, non una banca ma il gruppo dirigente di una banca che aveva perlomeno

la si salvava facendola acquistare da una banca cosiddetta buona. Che cosa abbiamo ottenuto? Molto spesso l'effetto contagio: la piccola mela marcia riusciva a far marcire l'intero cesto delle mele, i problemi. Con questa mancata vigilanza e mancata volontà di prendere decisioni nette ci è sembrato di aver salvato il sistema. lo abbiamo semplicemente coperto. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una situazione analoga e non vediamo di cosa ha bisogno la famiglia italiana, cioè di facilità di accesso al credito e di essere tutelata nel proprio risparmio. Lo avete visto, signori del Governo, che la gente sta scappando, sta correndo a recuperare i propri risparmi perché ha paura o non ha più fiducia nel sistema della gestione dei propri fondi da parte delle banche. Lo vedete cosa sta accadendo? Ancora una volta scegliete di stare dalla parte dei più forti.

Voi siete amici della finanza, non siete amici delle banche perché le banche, quando fanno bene il loro lavoro, a loro volta sono amiche dell'economia e sono amiche del tessuto familiare del nostro territorio. Bene: aiutate la finanza questo tetto fissato non al 18, non al 15, non al 20 ma al 17 per cento. E le eccedenze? Perché non pensate, fatelo con un prossimo provvedimento, ma soprattutto cercate di farvi un'idea e di dare un assetto organico a tutto il sistema. Ma perché non si possono risarcire tutti gli obbligazionisti che avevano affidato al sistema bancario i propri risparmi? Perché non andare davvero a determinare un'azione per cui

il sistema non può essere controllato? Ma di cosa stiamo parlando? Nella mia Provincia c'è una banca popolare che da sempre è stata uno degli elementi di successo, magari non controllabile e non gestibile.

Non possiamo votare la fiducia; non lo faremo purtroppo per una scelta del Governo di porre la fiducia, perché magari alcune parti del provvedimento avremmo pure potuto votarle, alcune condividere e altre contribuire a modificare. Ma voi ponete la fiducia. Ci chiedete se abbiamo fiducia in voi; vi rispondiamo: non abbiamo fiducia in voi, anche per come vi siete comportati con questo provvedimento. Ma siccome in dichiarazione di voto rappresento un Gruppo al cui interno vi sono dei colleghi che hanno una visione diversa, dico che per lo più il nostro Gruppo esprime sfiducia nei confronti della mozione posta dal Governo. *(Applausi dei

che prende in considerazione aspetti diversi: il rafforzamento delle strutture bancarie del nostro Paese con la trasformazione delle banche cooperative, il problema delle sofferenze bancarie, disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi, una più puntuale regolamentazione dei fondi di investimento alternativi, norme vincolanti per il calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente o di conto pagamento, una diversa regolazione dei rapporti con la Tesoreria centrale e la Cassa depositi e prestiti. problemi che, come si può vedere, non hanno la stessa valenza, ma riflettono un certo affastellamento di temi che forse non aiuta quella semplificazione legislativa da più parti evocata. Detto ciò, è bene separare e concentrarsi sugli aspetti più rilevanti. Il filo rosso è rappresentato dal rafforzamento del sistema bancario italiano, che oggi vive una stagione travagliata. è quello delle banche cooperative e delle sofferenze bancarie accumulate, per le quali si prevede la relativa cartolarizzazione assistita da garanzie dello Stato. Un tema, quest'ultimo, che ha fatto molto discutere, soprattutto in sede comunitaria, ove più volte è stato adombrato il pericolo di un aiuto di Stato, dimenticando quanto è avvenuto solo qualche anno fa, quando numerose banche europee sono state salvate grazie all'intervento diretto dello Stato sul capitale azionario delle medesime. La *ratio* del provvedimento mira a rafforzare l'architettura di sistema: scelta ineludibile. Le strutture finanziarie, non solo italiane, sono sottoposte a sollecitazioni crescenti. Un primo problema è dato da possibili *shock* simmetrici, che sono il prodotto della globalizzazione dei mercati. Lo si è visto chiaramente con il fallimento della Lehman Brothers. L'onda d'urto di quella crisi ha investito molti Paesi europei: Inghilterra e Germania, per non parlare di Spagna e Irlanda. In Italia ci siamo illusi che le nostre banche, per il fatto che non parlavano inglese (come si disse allora) ne fossero esenti: fu un errore. Il Governo non intervenne, sulla scia di analoghi interventi europei. Anzi, l'Italia finanziò il salvataggio delle banche degli altri Paesi, salvo poi dover prendere atto dell'accumularsi di sofferenze alle quali oggi si cerca di porre rimedio. Un secondo pericolo è rappresentato dagli *shock* asimmetrici. Questi ultimi sono conseguenza della peculiarità della situazione italiana; sono attribuibili, in altre parole, alla particolare configurazione del suo sistema economico. La crisi dell'economia reale in Italia è stata più forte che altrove; lo dimostra la forte caduta del reddito, quei 9 punti di differenza che ancora ci contraddistinguono rispetto alla media europea, un *gap* che recupereremo solo lentamente. Da un punto di vista territoriale, la crisi non è uniforme: molte aziende, specie al Nord, si sono riconvertite, mentre altre purtroppo, e sono in numero maggiore, stentano. La loro crisi si riflette sullo stato di salute delle banche minori, quando queste ultime sono troppo legate a quei territori. Nasce da qui l'esigenza di un loro rafforzamento patrimoniale. Si pensi a quanto avviene nel Veneto, in cui la Popolare di Vicenza e Veneto Banca vivono oggi una crisi profonda. Il problema delle banche popolari, troppo piccole e troppo legate ai singoli territori, va quindi affrontato alla radice, prevedendo forme di aggregazione che consentano, da un lato, di non disperdere le conoscenze specifiche dell'ambiente in cui operano e, dall'altro, di garantire la loro solidità patrimoniale, confluendo in un'organizzazione più solida. Questa è la scelta di fondo del decreto-legge al nostro esame. Si prevede infatti la nascita di un gruppo bancario, al quale le singole popolari devono confluire obbligatoriamente, la loro trasformazione in società per azioni, quando il loro capitale abbia una consistenza minima, che viene indicata in 200 milioni.

per cento del patrimonio netto), quale ristoro delle facilitazioni tributarie ottenute in passato, al pari di tutte le società cooperative. È quindi comprensibile che la loro trasformazione giuridica comporti anche un riallineamento sul piano tributario, nella presunzione che una parte del patrimonio netto posseduto sia stato anche il riflesso delle minori tasse pagate in passato. Nel nuovo regime giuridico avremo quindi un sistema bancario più solido. Tale passaggio potrà essere reso ancora più efficace

contro il 10,5 per cento delle altre banche. Perché è così importante risolvere questo problema? Innanzitutto per una ragione contingente. La loro presenza sui bilanci delle singole banche rischia di vanificare la politica della Banca centrale europea e gli sforzi di Mario Draghi per combattere la deflazione. Le banche, infatti, non riescono ad erogare credito alle strutture produttive finché i loro coefficienti patrimoniali sono intaccati dalla presenza di questo fardello, che non è poi così modesto, visto che si parla di 200 o di 80 miliardi di euro, a seconda che si consideri il lordo o il netto. Ripulire i bilanci delle singole banche diventa quindi essenziale per consentire loro di erogare credito, nel rispetto dei vincoli posti dalla sana e prudente gestione. Nel caso italiano, il fenomeno assume un peso ancor più rilevante a causa delle contraddizioni più generali della politica economica imposta soprattutto da Bruxelles. Il conflitto è quello tra una politica monetaria che punta ad un *target* d'inflazione del 2 per cento ed una politica di bilancio che è vincolata al rispetto del *fiscal compact*. Nel primo caso, infatti, si cerca di combattere la deflazione con misure non convenzionali. Nel secondo prevale l'ortodossia ed una stretta che nega, in radice, il tentativo di creare inflazione, alimentando al contrario una situazione tendenzialmente deflazionistica. Gli istituti di credito sono al centro di questa contraddizione. Hanno facilità di provvista, se non altro grazie alla Banca centrale europea, ma non hanno domanda di credito a causa del ristagno della domanda interna. Si trovano, pertanto, stretti in una morsa. I possibili margini di intermediazione si restringono. Il risultato finale è, inevitabilmente, la mancanza di utili d'esercizio o la crescita della sofferenze, a causa della crisi dell'economia reale. Il decreto-legge al nostro esame cerca, per quanto possibile, di farsi carico di questa contraddizione, dando ossigeno agli istituti di credito, consentendo loro di sbarazzarsi, con la cartolarizzazione assistita da garanzia statale, delle sofferenze a bilancio. Ma è evidente che la soluzione fisiologica sia altrove. Occorre, in altre parole, riconciliare politica di bilancio e politica monetaria per indirizzarle, entrambe, verso un unico obiettivo. Finché ciò non avverrà, sarà difficile che il problema possa trovare una soluzione definitiva. Per i motivi esposti

Signora Presidente, la riforma delle banche di credito cooperativo intende proseguire l'opera di riassetto e di innovazione del sistema creditizio italiano, già intrapresa con la riforma delle banche popolari. Com'è noto, l'esercizio dell'attività bancaria in forma di credito cooperativo in futuro è consentito esclusivamente alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. aderiscano a tale gruppo si prevede un meccanismo di *way out* fedele al modello cooperativo. I requisiti introdotti con la presente riforma favoriscono l'accesso al mercato dei capitali, nonché la patrimonializzazione della capogruppo e degli istituti aderenti. Così si determinano le condizioni per una loro competitività ed efficienza. Si introducono, dunque, regole innovative nella gestione del risparmio che consentano di favorire il credito alle imprese e di prevenire o gestire meglio eventuali situazioni di crisi. Ciò avviene con attenzione alle realtà virtuose presenti nel sistema del credito cooperativo e al loro rapporto con il territorio, dunque salvaguardando anche le loro finalità mutualistiche. Nell'ambito della riforma il punto decisivo per noi autonomisti è stato senz'altro il riconoscimento del diritto di costituire una *holding* autonoma con sede in provincia di Bolzano, a condizione che le banche partecipanti e la banca capofila operino esclusivamente nel territorio provinciale e abbiano sede nel medesimo territorio. Analoghe norme e possibilità sono previste per la Provincia autonoma di Trento. L'intesa raggiunta attraverso una proposta di modifica, che abbiamo definito con il Governo e con la maggioranza, salvaguarda quindi l'autonomia delle casse rurali sudtirolesi. È stato quindi riconosciuta la particolarità del sistema Raiffeisen, oggi vigente. Le casse Raiffeisen svolgono già oggi un ruolo importantissimo per l'economia locale. Inoltre queste casse hanno anticipato il sistema nazionale con la creazione della Cassa centrale, una capigruppo in forma di SpA che opera da tanti anni nella nostra Provincia e che coordina e rafforza le singole casse aderenti. Questo modello di successo, la cui solidità è stata riconosciuta ed apprezzata anche dalla Banca d'Italia, viene così salvaguardato. Ora spetterà alla Banca d'Italia definire i requisiti relativi al patrimonio netto della capogruppo ed alla dimensione del gruppo, tenendo evidentemente conto della limitata delimitazione territoriale. Tale deroga, introdotta in sede di conversione del decreto-legge, elimina dalla riforma vincoli e parametri che avrebbero impedito al sistema Raiffeisen di continuare ad operare e salvaguarda anche le competenze legislative e statutarie della Regione Trentino-Alto Adige in ordine al mondo della cooperazione. Dunque, si tratta di una soluzione che non penalizza, ma - all'opposto - premia i criteri di prudente gestione ed efficace organizzazione del credito, che sono - anche questi - gli obiettivi della riforma

grande attenzione e sensibilità ai problemi posti. In questo senso, colgo l'occasione per ringraziare il vice ministro Morando per l'ottimo e faticoso lavoro

a favore della questione di fiducia posta dal Governo.

quest'Assemblea e tutto il Parlamento. Credo che una riforma organica del sistema delle banche di credito cooperativo attuata con decreto-legge non sia certamente il modo migliore per affrontare un problema così complesso.

forse la prova di quale sia ormai il grado di rapporto tra la funzione legislativa e quella esecutiva.

(un importo considerevole se si pensa che, fino all'emanazione del provvedimento, bastavano 2 milioni di euro per costituire una nuova banca). Le piccole, o quelle che non ritengono di doversi fondere con altri istituti, sono costrette, volenti o nolenti, a sottoporsi a un ombrello di controllo a una *holding* stabilita per legge. Inoltre, per quelle stesse BCC che dovessero decidere di esercitare il *way out* è prevista la trasformazione forzata in società per azioni ed il versamento di una quota, a titolo d'imposta, pari al 20 per cento del patrimonio netto, con il serio rischio di esporre un intero sistema ed un patrimonio costruiti da generazioni di soci a tentazioni opportuniste da parte di chi ne potrebbe disporre senza quegli stessi vincoli che ne hanno determinato nel tempo l'accantonamento. Questa possibilità renderà evidentemente conveniente per i soci la trasformazione rendendo distribuibili ai soci, divenuti azionisti, ingenti somme precedentemente indivisibili, permettendo loro di realizzare enormi plusvalenze. Alla fine di questa strada non riteniamo ci sia un credito cooperativo più forte; c'è un credito cooperativo demolito a favore di un sistema privatistico di capitale qual è quello delle società per azioni. Il credito non verrà più erogato secondo le regole cooperative, cioè privilegiando i propri soci per almeno il 51 per cento; le SpA potranno essere cedute, e quindi anche penalizzando i territori in cui sono insediate, e si aprirà all'ingresso di gruppi di natura privatistica. Le regole dovrebbero inoltre essere uguali per tutti: se si riconosce il diritto di trasformarsi in SpA per non sottoporsi ad un vincolo, anche pesante, di vigilanza interna, che può arrivare anche fino al commissariamento, dovrebbe essere riconosciuto a tutti gli istituti. istituti. Non si comprende poi perché, alla luce della riforma, debba essere consentito il passaggio da banca di credito cooperativo, ossia da una banca cooperativa a mutualità prevalente, ad ordinaria società commerciale, con relativa possibilità di affrancamento, e debba essere invece esclusa tale possibilità se la società risultante è costituita in forma di banca popolare, banca sempre cooperativa, ma a mutualità non prevalente. Rimangono ancora non chiare le modalità con cui le BCC possono costituire il capitale della *holding* perché non si precisa se debba essere capitalizzata per contanti o attraverso il conferimento di *asset*. *asset*. La previsione che permette alla *holding* di commissariare i livelli di governo delle singole BCC non più in casi motivati ed eccezionali, come previsto in origine dal testo presentato dal Governo, ma semplicemente adducendo una motivazione, non prevede come contrappeso che il contratto di coesione garantisca alle banche aderenti al gruppo un grado elastico di autonomia rapportato alla capacità di ognuna di esse di mantenere solida la propria situazione patrimoniale e redditizia, la propria attività corrente, facendo in tal modo perdere loro progressivamente autonomia trasformando le BCC aderenti al gruppo cooperativo in filiali di una banca unica o, peggio, dando il via ad una banca che può diventare proprietà anche di fondi esteri e che può commissariare liberamente tutte le banche sottostanti. Si crea, quindi, un modello ibrido che, oltre a non riuscire a replicare i modelli presenti in altre Nazioni europee per evidenti disparità dimensionali, fa perdere tutte quelle peculiarità della cooperazione nel settore creditizio, nel settore creditizio, tese a valorizzare le specificità locali, culturali e socio-economiche dei diversi territori italiani. In sostanza, si crea un sistema con il quale si facilita il commissariamento delle BCC aderenti al gruppo da parte della *holding*, si spingono le piccole BCC a fondersi con le grandi per poter esercitare la *way out*; si consente alle grandi BCC di derogare a quella mutualità prevalente che fino ad oggi ha favorito il credito a PMI e famiglie. Con questa riforma si mette in moto un meccanismo che di virtuoso non ha nulla. Mentre si dice di voler fare una *holding* unica a tutela del credito cooperativo e, quindi, anche della sua prospettiva futura, in realtà si vara una legge che andrebbe chiamata in modo completamente diverso, perché il suo unico effetto è quello di spingere le banche di credito cooperativo ad aggregarsi, a raggiungere il livello minimo di patrimonio netto e a trasformarsi in SpA.

si riverbera nella previsione contenuta nel provvedimento secondo cui il MEF si è riservato la possibilità di cambiare la legge, con proprio decreto, modificando la percentuale di possesso azionario del nuovo grande gruppo cooperativo, che il decreto-legge oggi prevede al 51 per cento nelle mani delle singole BCC che lo compongono. cento è una base minima per offrire una garanzia di autonomia alle banche cooperative che compongono la *holding* e costituisce quindi una barriera allo snaturamento delle finalità cooperativistiche. La possibilità affidata al MEF di modificare con decreto tale percentuale, abbassandola al 40, al 30 o addirittura fino al 10 per cento, apre oggettivamente la strada alla possibilità concreta di privatizzazione del gruppo comprendente tutte le BCC italiane, che potrebbe così trasformarsi in SpA nelle mani di altre banche di maggiori dimensioni dimensioni o, peggio ancora, di fondi esteri. Ciò che si riverbera in questo aspetto del decreto-legge è la paura e l'ossessione europea di un'Italia che possa contagiare con la propria, presunta, instabilità Il Governo offre puntualmente una soluzione di passiva acquiescenza in tal senso, senza minimamente tutelare l'interesse del Paese e della nostra economia, che fonda le sue basi su una diffusa e robusta rete di piccole e medie imprese, che trova e ha trovato, in larga parte del territorio, una efficace e fondamentale sponda nel tessuto del credito cooperativo

Signora Presidente, signor vice Ministro, ho riflettuto se fare o no questa dichiarazione di voto, perché nel decreto‑legge in esame viene introdotta una norma che ritengo sbagliata e che può costituire un grave precedente per la cooperazione italiana. Se l'*iter* legislativo fosse partito dal Senato, quella norma probabilmente sarebbe stata ulteriormente ridimensionata, se non addirittura cassata. Quando si riduce il Senato a dire solo un «sì» o un «no», non solo si riduce la funzione legislativa, ma si rende la democrazia mediocre. Con altrettanta onestà intellettuale riconosco che l'impianto del decreto-legge, nei suoi vari titoli e con le modifiche importanti e le integrazioni altrettanto importanti avvenute in Commissione finanze alla Camera anche grazie al lavoro del vice ministro Morando, che ringrazio - è convincente e utile per il Paese. Non siamo un Gruppo guidato da un'ideologia, non siamo un Gruppo manicheo o un Gruppo che fa demagogia e quindi non riteniamo che la crisi abbia un solo responsabile. La crisi che ha attraversato il Paese ha genitori sparsi in tutti i settori dell'economia e delle istituzioni. Dunque, le banche non sono affatto esenti da critiche, ma rimangono per noi degli intermediari essenziali per il sostegno alla ripresa economica. quindi che la magistratura, la Banca d'Italia e gli organi statutari delle stesse banche perseguano, nel rispetto della legge, gli amministratori disonesti e quelli incapaci degli istituti di credito, alcuni anche importanti, in grave crisi o andati in *default*. Riconosciamo però che negli ultimi sette anni il sistema bancario italiano ha affrontato prima una crisi finanziaria, che veniva da Oltreoceano, poi una crisi dei debiti sovrani e infine una crisi dell'economia reale, senza scaricare i costi sui contribuenti italiani.

(per non parlare dell'Irlanda e della Grecia). I molti casi di insolvenza si sono tradotti nelle banche in un aumento considerevole dei crediti deteriorati, e poiché l'Italia ha bisogno di intermediari finanziari forti sul piano patrimoniale, capaci quindi di dare credito, cioè fiato, a imprese e famiglie, l'intervento del Governo diventa - ed è stato - importante e necessario. Come ha ricordato nella sua ragionata e convincente replica il vice ministro Morando, il decreto-legge si muove nella direzione giusta sia quando riforma il credito cooperativo sia quando costruisce un mercato delle sofferenze bancarie con la concessione delle garanzie dello Stato alle *tranche senior* delle cartolarizzazioni sia anche quando interviene in materia tributaria con il pacchetto fiscale. È stato detto che la riforma delle banche di credito cooperativo stronca l'unica presenza davvero localistica e partecipata nel mondo del credito bancario. Se così fosse, io per primo inviterei il Senato a votare contro il Governo. Ragioniamo: le BCC in Italia sono 360 e sono nate centotrenta

Le BCC attraversano tre secoli con tre riforme, compresa questa. Nascono per rispondere ai bisogni delle popolazioni rurali contro gli usurai. Nel 1937 si aprono al mondo artigianale e nel 1993 si aprono a tutte le categorie, con una pratica al dettaglio, facendo *retail*. Anche con le importanti riforme del 1937 e del 1993 si disse che le banche di credito cooperativo, allora casse rurali, sarebbero diventate un'altra cosa. Sarebbe finita in esse finita in esse la democrazia economica e la partecipazione e sarebbero state spazzate via dalla competizione. Sarebbero state omologate alle altre banche. Eppure, mentre il numero delle BCC scende, con queste riforme si espande la presenza sul territorio, tanto da ricoprire 2.700 Comuni, e negli ultimi vent'anni i soci salgono in maniera esponenziale. Grazie alla coerente applicazione delle regole della buona cooperazione, la patrimonializzazione delle BCC è stata superiore al resto del sistema: più 20 per cento, pari a 20,5 miliardi di questi tempi. Ma le BCC, come le cooperative, non sono di un altro mondo. In un mercato in continua evoluzione e con una maggiore concorrenza, le cooperative devono sapersi modellare alle logiche del mercato. Il problema è che non perdano l'anima: senza vendere l'anima. In alcuni settori di tradizionale insediamento cooperativo, come l'agricoltura, il consumo e appunto il credito, è finito il tempo delle cooperative solitarie, delle cooperative atomistiche, non integrate in un gruppo o in un consorzio cooperativo o in una filiera cooperativa. La crisi economica prolungata espone le banche di credito cooperativo che fanno *retail*, e le espone di molto. di molto. I soci persone fisiche in passato si sono messi insieme per fare una cooperativa, per fare una BCC contro gli usurai. Oggi anche le cooperative si devono mettere insieme e fare cooperazione tra cooperative, per difendere i valori di democrazia economica, di partecipazione dal basso, di difesa dei più deboli nell'economia e, soprattutto, per svolgere fino in fondo la loro missione.

in Spagna e nella stessa Olanda, che è stata il punto di riferimento con un gruppo già integrato intorno a Rabobank e che ancor più si integra oggi. Ci sono e ci saranno Se le cooperative di credito italiano rimanessero così come sono, inizierebbe il declino e alcuni segnali, alcuni scricchiolii già oggi si avvertono. Dunque, la riforma che oggi votiamo favorirà la nascita di un gruppo bancario con una solida capogruppo, il cui capitale maggioritario è in mano alle BCC; un gruppo che si fonda sul protagonismo della singola banca di credito cooperativo, che rimane intestataria della licenza bancaria e dove rimane intatta la pratica della mutualità e della partecipazione cooperativa. A differenza di quanto avviene in Europa, è stata introdotta la gradazione dei poteri della capogruppo in relazione al grado di meritevolezza della singola BCC. I poteri della capogruppo saranno proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti. Ecco perché questa è una grande riforma. Bisogna riconoscere alla Federcasse di essersi autoriformata, di avere proposto un progetto, e riconoscere che il Governo ha di fatto validato questa riforma. Dunque, alle preoccupazioni che con questo decreto-legge si imbocca la strada dell'omologazione forzata del credito cooperativo al gigantismo bancario la nostra risposta è no: questa è una vera, autentica, riforma Il Senato, quindi, scrive oggi una pagina storica, una pagina di rafforzamento, di crescita e di sviluppo del mondo delle banche di credito cooperativo, senza che queste banche perdano l'anima.

che la Camera ha tentato di ridurre, ma che c'è, è visibile ed è foriera di problemi. L'introduzione di una via d'uscita, la cosiddetta *way out*, risponde all'esigenza particolare - diciamocelo pure - di alcuni cooperatori da quartierino; rischia di inficiare il disegno strategico spezzettando il sistema; introduce un *virus* nella prassi e nei principi cooperativi. La *way out* non è un'invenzione di oggi.

chi dice che l*a way* *out* risponde al dettato costituzionale dell'articolo 41 della Costituzione, di rispettare, cioè, l'attività imprenditoriale, rispondo, però, che la medesima osservazione non è stata tenuta in considerazione quando si sono trasformate in modo coatto - anche con il mio voto convinto - le banche popolari in SpA. La *way out* genererà delle cooperative geneticamente modificate, degli OGM cooperativi, delle cooperative che si spogliano della loro missione e della loro storia e che il giorno dopo si metteranno alla ricerca - sempre con quegli stessi camaleonti - di un'uscita dal blocco delle riserve indivisibili e delle indisponibilità del patrimonio per trasformare i cooperatori in azionisti. Concludendo, pesa pesa di più la macchia o il progetto? Pesa indubbiamente di più la costruzione di un progetto strutturale per la finanza del Paese e per le banche di credito cooperativo. Per questo dichiaro il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge e alla fiducia al Governo.

Come ribadito ieri, ci troviamo oggi in quest'Aula a parlare di banche e anche oggi lei e il suo Governo avete posto la fiducia. Certo che avete un bel coraggio: questo nessuno lo può negare. Lei e il suo Governo siete coinvolti in diversi scandali e indagini e continuate a dire che va tutto bene. non ci meravigliamo del suo atteggiamento, ma ci stupisce il comportamento dei parlamentari che sostengono il suo Governo senza sapere cosa gli farà votare di volta in volta. A regola, in questo maxiemendamento non dovrebbero sorgere nuove marchette per i suoi amichetti perché è già tutto molto chiaro. Lei, con tutto il suo Governo, rappresenta solo gli interessi delle *lobby*, una piccola cerchia di persone che detengono, da sole, quasi tutta la ricchezza del pianeta e continuano a volerne sempre di più a danno dei cittadini che lavorano o che vorrebbero lavorare dignitosamente. Vorrei ricordarle che nonostante non abbia mai ricevuto l'avallo del popolo italiano per il suo incarico, lei dovrebbe rappresentare e difendere gli interessi dei cittadini italiani. È persino chiaro il messaggio che il senatore a vita Mario Monti le ha lanciato in quest'Aula. Sembrava voler dire: stai attento a come ti comporti, sei nel mirino, non denigrare troppo l'Europa perché potrebbe esserti fatale, metaforicamente parlando. Infatti, lei ha recepito il messaggio ed è corso subito ai ripari: provvedimento a favore delle grandi banche per arrivare, dopo l'unione monetaria, all'unione bancaria europea con l'obiettivo di un Ministero delle finanze europeo che controllerà e gestirà l'economia dell'Unione europea. Sarà ben felice il senatore Napolitano: il nuovo ordine mondiale sta per essere portato a compimento. Questa manovra, con tutte le altre che andate presentando e farneticando in TV o nei salotti non porterà nessun beneficio alle persone e all'economia reale. Non è vero che queste riforme consentiranno alle banche di dare credito alle piccole imprese o alle famiglie in difficoltà. È una bugia. Il sistema bancario italiano ha bisogno di amministratori sani e di veri controlli. Bisogna dividere le banche d'affari dalle banche commerciali. Bisogna stabilire regole e sanzioni per chi truffa i risparmiatori,

oppure a chi vanta amicizie che contano. Ne sono la riprova le sofferenze bancarie che vanno imputate ai grandi gruppi industriali o alle imprese costruttrici che hanno fatto investimenti sbagliati di cui già si conosceva il risultato. Ma i favori agli amici portano voti, i voti portano potere e il potere porta soldi. Quando farà un decreto-legge per istituire il politometro? I cittadini quando potranno sapere se un politico, dopo anni di carriera, ha aumentato il suo patrimonio in modo spropositato? Dimenticavo, il suo obiettivo non è il benessere dei suoi concittadini. Ma faceva tanto comodo a qualcuno: vedi speculazioni accadute. Poi nuove cartolarizzazioni, ossia finanza creativa e speculativa su crediti deteriorati e di difficile di difficile incasso, con possibilità per le banche di detrarre le perdite sui crediti in un solo anno e non più in Poi abbiamo l'entrata in vigore del *bail in*, dove i risparmiatori, quelli che hanno un conto corrente e che non hanno fatto nessun investimento, potrebbero essere chiamati a rispondere delle perdite bancarie.

Poi arriviamo al decreto legislativo dove stabilite che il finanziatore (di solito la banca) possa entrare direttamente in possesso del bene posto in garanzia senza la verifica di un giudice terzo. li ho sicuramente dimenticati. Oggi, invece, con questo decreto-legge reinserite l'anatocismo bancario: la maturazione di interessi sugli interessi, come fanno gli usurai, e nuove cartolarizzazioni coperte dallo Stato, con i soldi che erano destinati a garantire i debiti che la pubblica amministrazione non ha ancora pagato ai suoi creditori. Questo sempre per l'economia reale? questi sarebbero provvedimenti a favore dei cittadini e delle piccole e medie imprese, a favore dell'economia? State rendendo questo Paese schiavo: lavoratori precari con case precarie. Vi fa comodo governare persone sempre sotto ricatto per fame. Utilizzate il ricatto dei posti di lavoro anche per la campagna referendaria del 17 del 17 aprile contro le trivelle, senza tenere conto dei danni che state procurando all'ambiente e alle persone, con notevoli costi per la sanità e le bonifiche. Vergogna. Non so quanti di voi conoscano persone con stipendi di 800-1.000 euro al mese, con i quali devono pagare l'affitto o il mutuo, far mangiare la famiglia, mandare i figli alla scuola dell'obbligo; per non parlare delle scuole superiori e dell'università. In due anni del suo Governo, io e tutti i cittadini non abbiamo mai visto un provvedimento a nostro favore. Manca pure un sistema di garanzia e assistenza per chi frequenta la scuola dell'obbligo. Ma questo non interessa a nessuno. Per voi meglio un Paese schiavo e ignorante. Vergogna. Le famiglie con più figli ogni anno devono comprare libri scolastici nuovi anche per la scuola dell'obbligo. Lo studio non è solo obbligatorio, ma è un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Vergogna. Sarei curiosa di vedere ognuno di voi vivere nelle stesse condizioni anche solo per una settimana; provare il dolore di dover dire al proprio figlio: non posso comprarti neppure un ghiacciolo perché non ho i soldi. A noi cittadini servono atti concreti che ci consentano di vivere serenamente e dignitosamente, come

Avete una visione del mondo e dell'Italia come i cavalli quando hanno i paraocchi. Sapete andare solo avanti senza rendervi conto di ciò che accade intorno. Il Paese ha bisogno di un Governo diverso, ha bisogno di persone oneste e con le mani libere. E, fino a quando non ci sarà un Governo a 5 Stelle, continueremo ad urlare la nostra indignazione e il nostro convinto no a questi infami provvedimenti a danno del buon nome dell'Italia e del benessere dei cittadini. Colgo inoltre l'occasione per ricordare a tutti che abbiamo presentato una mozione di sfiducia a questo Governo e che ne attendiamo la calendarizzazione al più presto. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge in esame interviene sulla regolamentazione delle banche di credito cooperativo, modificando ampiamente il testo unico in materia bancaria e creditizia. Esso precisa inoltre altri temi, che riguardano la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Preliminarmente, va sottolineato che, nonostante Federcasse (la federazione che raggruppa le ex casse rurali e artigiane) abbia condiviso questa riforma, molti sono ancora i dubbi e i timori espressi dalle tante realtà del credito territoriale, che sentono minacciata la propria autonomia. Infatti molte di queste piccole realtà vedono minato il fondamento e l'essenza stessa dei piccoli istituti di credito, che, nati per iniziativa dei territori di riferimento, lavorano a supporto quasi esclusivo di queste realtà, creando con questo intervento un danno al sistema di credito italiano. La trasformazione in nuovi soggetti delle banche di credito cooperativo non porterà a un rafforzamento del settore bancario, né garantirà che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese, favorendo quindi la disponibilità di servizi migliori a prezzi più contenuti. Al contrario, anche quella parte di credito sinora dedicata al territorio potrebbe essere relegata nei più rigidi parametri dell'assegnazione del merito di credito, seguita dalle grandi banche o dai grandi gruppi bancari, con criteri standardizzati su tutto il territorio nazionale. La disposizione si scontra, con tutta evidenza, con i principi costituzionali di libertà di impresa, prevedendo la trasformazione in società cooperative per azioni che potranno esercitare l'attività bancaria solo se appartenenti a un gruppo bancario cooperativo. Se consideriamo i dati sul credito nel nostro Paese, l'insieme delle banche di credito cooperativo ha registrato un aumento dei crediti erogati alla clientela. Al contrario, le banche aventi natura di società per azioni hanno ridotto l'ammontare dei prestiti e persino i grandi gruppi bancari esteri presenti nel nostro Paese hanno registrato un segno negativo nell'erogato. La gran parte dei crediti delle banche di credito cooperativo sono stati deliberati a favore piccolissime, piccole e medie imprese. Se non vi fosse stata questa grande massa di crediti, molte imprese sarebbero andate in crisi, determinando quindi certamente un aumento del numero di persone senza posto di lavoro. Vorrei anche sottolineare che, nonostante le sofferenze, le piccole banche territoriali sono riuscite a mantenere un alto livello di patrimonializzazione. In tal senso, va considerato che l'indice con cui si misura la patrimonializzazione (CET1) delle banche di credito cooperativo nel 2014

Le BCC vantano un patrimonio consolidato di 20,2 miliardi di euro e rappresentano la terza realtà bancaria italiana. Ma al contempo le BCC, presenti con 371 istituti, hanno una presenza di prossimità rilevante, con 4.450 sportelli in 2.697 Comuni In particolare, le BCC hanno destinato il 96 per cento dei finanziamenti, pari a 92 miliardi nel 2014, alle imprese e alle famiglie. Tradotto in soldoni, hanno consentito a una famiglia su cinque di accedere a un mutuo per l'acquisto della casa ed hanno consentito alle imprese micro, piccole e medie che sono l'ossatura del nostro sistema produttivo, di investire nella propria attività, salvaguardando - come ho detto prima - posti di lavoro. La spinta al credito è dimostrata dall'accettazione dell'84,8 per cento dei finanziamenti richiesti, rispetto al 75,3 per cento delle altre banche. Va considerato inoltre che la prossimità la conoscenza del territorio di norma riducono il rischio del prestito stesso e in particolare che le BCC hanno registrato un tasso di sofferenze nei prestiti alle imprese pari al 21,6 per cento, rispetto al 33,7 per cento delle altre banche. Le BCC, in quanto banche di prossimità, hanno seguito sino alla fine i propri creditori e non li hanno abbandonati al proprio destino, come spesso hanno fatto le grandi banche non radicate territorialmente. Esse sono state, inoltre, protette dalla bassa esposizione alla volatilità della raccolta all'ingrosso e dal peso limitato degli investimenti finanziari. Insomma, hanno continuato a curare la loro clientela di elezione, come ho già detto, le imprese di minori dimensioni e le famiglie, avendo il vantaggio di disporre di informazioni, anche qualitative, che hanno reso più efficaci le politiche di erogazione del credito. Si sono così in parte attutite per il sistema economico le conseguenze della diminuzione dell'offerta di credito da parte delle banche maggiori. Proprio nel periodo di crisi, le banche del territorio, pur faticando a salvaguardare la loro stabilità di fronte alla pressante richiesta che viene dalle comunità di riferimento, hanno agito da veri e propri ammortizzatori degli *shock* economici. di credito cooperativo contengono in sé il carattere della mutualità, ovunque prevista dai loro statuti, tutelata dalla Costituzione. Il carattere della mutualità trova riferimento, innanzitutto nella valutazione del merito di credito che le banche di credito cooperativo concretizzano nei confronti di 1.230.308 soci, della clientela e del territorio di riferimento. È presente una mutualità a favore dei soci, ma sopratutto una mutualità indirizzata a favore delle economie locali servite dalla banca, come provato dalle clausole statutarie di tutte le banche di credito cooperativo. Vale la pena ricordare che ammontano a 755 milioni i microcrediti erogati dalle banche di credito cooperativo, in larghissima parte destinati a combattere situazioni di fragilità economica e sociale.

E questo a riprova del carattere prettamente mutualistico delle strutture societarie cooperative di queste banche nei confronti dei territori. Un aspetto su cui vorrei fare una riflessione, sollevato anche da Federcasse, è che questo decreto-legge lederebbe la Carta costituzionale all'articolo 41, perché rischia di imporre un limite al libero sviluppo della forma cooperativa nel settore bancario. Questo provvedimento è un intervento a gamba tesa sul credito cooperativo, andando a minare anche i principi che incoraggiano e tutelano il risparmio, laddove le banche territoriali saranno sostanzialmente costrette a convergere nell'unico gruppo bancario centralizzato. Va rilevato ancora una volta che, anche in questo caso, la prossimità territoriale delle banche equivale a un maggior controllo da parte dei correntisti e alla conseguente maggiore tutela dell'integrità del risparmio stesso. Il decreto-legge contiene altre norme che ci vedono fortemente contrari che riguardano le disposizioni per la cartolarizzazione e gestione delle sofferenze, sui quali i miei colleghi di Forza Italia sono intervenuti in discussione generale e che quindi qui voglio solo ricordare come titolo. Per questa ragione, dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia perché questo provvedimento mortifica quelle realtà del Paese che di fatto stanno reagendo alla crisi; ma in più dimostra, ancora una volta, la mancanza di strategia di questo Governo e l'incapacità di dare risposta ai problemi reali degli italiani. *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, vice ministro Morando, gli interventi del relatore e dei colleghi del Partito Democratico Fornaro e Marino mi facilitano questa dichiarazione di voto e quindi mi limiterò solo a considerazioni politiche di carattere generale. Tra l'altro, il Vice Ministro ha già spiegato, oltre alle questioni di merito, anche le questioni di metodo per cui il Governo ha scelto la strada del decreto-legge.

più di 900 casse rurali e nei diversi passaggi costituzionali e legislativi del Novecento hanno mantenuto sempre il fondamento della mutualità, fondato sul principio della reciprocità in una visione di lungo periodo e intergenerazionale. Nei lunghi anni della crisi, il PIL italiano ha perso il 9 per cento, gli investimenti fissi lordi si sono ridotti di circa il 30 per cento, la produzione industriale ha registrato un calo del 25 per cento e forti sono state le ricadute sul sistema creditizio, con un incremento delle sofferenze, delle perdite su crediti e con riflessi negativi sulla redditività del settore, con inevitabili effetti sul sistema produttivo, in particolar modo sulle piccole e piccolissime imprese. In questo contesto, le banche di credito cooperativo hanno svolto un ruolo fondamentale nei confronti di interi settori produttivi in difficoltà, in particolar modo quelli rivolti al mercato interno. La lunga recessione è stata uno spartiacque per l'economia occidentale e per il sistema bancario europeo, in particolare. La crisi ha spinto verso il compimento dell'unione bancaria europea, accompagnato da nuove e più stringenti regole di *governance* ed erogazione del credito. In questo nuovo contesto, alcuni Paesi hanno ritenuto di intervenire direttamente con ingenti iniezioni di liquidità per sostenere il sistema; altri, come l'Italia, hanno scelto di adoperare un'altra leva, quale quella di interventi legislativi sistemici senza impegnare risorse pubbliche. Se avessimo fatto come Germania, Francia e Spagna, avremmo dovuto investire 130 miliardi di euro, cosa improponibile Tutto ciò porta l'intera regolamentazione italiana ed europea a spingere in direzione di un rafforzamento patrimoniale del sistema bancario, al fine di aumentare la capacità di risposta, con il sistema delle banche di credito che però continua ad esprimere una grande vitalità per effetto soprattutto dell'ampia e diffusa articolazione territoriale, come è stato detto da più colleghi. una riforma necessaria, perché appare pressoché impossibile fare banca di prossimità e mutualistica in solitudine (mi permetterei di dire

come si è ribadito un anno fa in occasione della riforma delle banche popolari. Così è stato. La prima sfida è partita da qui e la prima sfida vinta è stata questa: un ampio dibattito interno, proposte concrete, verifica della conformità con le sempre più omologanti norme dell'Unione bancaria e dei principi contabili internazionali, confronto serrato a livello politico e tecnico con la Banca d'Italia e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

la libertà d'impresa fondata sulle capacità e sulla responsabilità; l'autoaiuto; la mutualità; la sussidiarietà; la partecipazione e il protagonismo delle comunità e dei territori; il controllo democratico da parte dei soci. L'impianto essenziale era stato accolto già nel decreto-legge emanato dal Governo il 10 febbraio scorso, poi arricchito e reso più equilibrato dal dibattito politico e parlamentare, recepito dal testo approvato dalla Camera dei deputati con le importanti modifiche apportate in merito alla nuova *way out,* alle riserve indivisibili e, in particolare, alle cartolarizzazioni. Oggi si può dire che quei punti dell'autoriforma sono stati tutti sostanzialmente accolti. Non lo dico io, ma lo sostengono gli stessi attori dell'autoriforma e chi non è condizionato da strumentalità politica, ed è quello che ci interessa. Ne è nato un modello giuridico che si ispira ad un approccio culturale ben preciso, sintetizzato in quei punti sopra richiamati, che vedrà la nascita di una realtà nuova sotto molti profili:

resterà una cooperativa a mutualità prevalente (ovvero erogherà il credito prevalentemente ai soci), con una propria licenza bancaria e un proprio consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea dei soci. cento almeno degli utili dovrà andare a riserva indivisibile. Il 95 per cento del totale dei crediti andrà erogato a famiglie e imprese del territorio e il risparmio della comunità verrà reinvestito nella comunità stessa. cooperativo sarà legata al gruppo tramite un sistema di cosiddette garanzie incrociate (forma di solidarietà che si combina ai concetti di responsabilità e di condivisione). Si conserverà la propria autonomia graduata sulla base della propria capacità. Meno risulterà rischiosa, secondo parametri oggettivamente misurabili, e maggiori saranno gli spazi di autonomia nella pianificazione e nella gestione della specifica missione nel territorio. una forma di coesione integrata, del tutto originale, nel mondo imprenditoriale italiano e, probabilmente, anche in quello europeo che fa di questa riforma un passaggio virtuoso fondamentale e imprescindibile nel processo riformatore del nostro Paese. In conclusione, la soluzione ricercata sta nella capacità di sviluppare, da parte dell'intero sistema, un marcato orientamento al mercato, una pratica trasparente della concorrenza e un preciso potenziamento strategico. In tal senso, la sfida è prima di tutto aziendale, ovvero visione e managerialità, soddisfazione del cliente e innovazione nei servizi. Tali obiettivi sono realizzabili se le imprese restano solide e patrimonializzate, condizione necessaria ed imprescindibile per una buona politica di investimenti.

Stefani).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Stefani.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2298, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, nel testo approvato dalla Camera dei deputati,

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito a maggioranza che martedì 19 aprile, alle ore 16,30, saranno discusse le mozioni di sfiducia al Governo nn. 551 e 554, presentate rispettivamente dai Gruppi Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega Nord, Conservatori e Riformisti. Conformemente alla prassi, i tempi del dibattito saranno quelli normalmente riservati alle mozioni e per ciascuna mozione di sfiducia avrà luogo un'autonoma votazione per appello nominale.

allo scandalo trivellopoli: uno scandalo che ha costretto il ministro dello sviluppo economico Guidi a dimettersi; uno scandalo ampiamente anticipato il 18 dicembre 2014 in quest'Aula dal senatore Cioffi, quando ha denunciato l'inserimento, all'interno del maxiemendamento, di un emendamento del Governo che andava a gli interessi della Total. Uno scandalo ampiamente denunciato da tutti gli organi di stampa che riportano le intercettazioni che coinvolgono questo Governo e

Un filone d'inchiesta che va ad interessare anche il Ministro della Difesa, uno scandalo che riguarda la flotta navale e che coinvolge tutto il Governo in quanto nel maxiemendamento presentato in quest'Aula dalla ministra Boschi è stato chiaramente inserito quell'emendamento voluto dalla ex ministra Guidi e dal suo compagno Gemelli. Uno scandalo chiaramente collegato agli interessi petroliferi di questo Governo, uno scandalo che riguarda tutto tutto quello che sta avvenendo, come i disastri ambientali che questa politica del fossile ha provocato nei nostri territori, che questa politica del fossile, questa politica

tutti i cittadini e tutte le famiglie italiane che in questo momento soffrono per i danni ambientali che sono stati causati da queste aziende e dal vostro comitato d'affari.

con onorabilità, dovrebbe percorrere il suo tragitto con onore, nel rispetto dei cittadini italiani e del territorio italiano. Quindi, se proprio non ha nulla da temere, è assurdo la maggioranza voglia spostare la discussione al giorno 19. I tempi utili ci sono. La calendarizzazione delle mozioni può avvenire immediatamente già da sabato, già da lunedì, già da martedì. il Movimento 5 Stelle non accetta assolutamente la volontà di questo Governo di rimandare il problema e non venire a rispondere in quest'Aula al Parlamento italiano, ma soprattutto di non venire a rispondere in quest'Aula ai cittadini della Basilicata, ai cittadini della Sicilia e a tutti i cittadini che in questo momento, in Italia, soffrono

ciò che pensa di questo Governo e cioè che se ne deve andare a casa immediatamente perché qui gli interessi dei cittadini sono l'ultima cosa di cui ci si occupa.

Signor Presidente, come abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo, noi chiediamo che le mozioni di sfiducia presentate da Forza Italia, Lega, Conservatori e Riformisti e Movimento 5 Stelle vengano calendarizzare e vengano trattate all'inizio dei lavori della prossima settimana, cioè martedì.

il signor Renzi ha dimostrato di fregarsene delle istituzioni, di fregarsene di tutto quello che viene chiesto dal Paese. Oggi come oggi, il 54 per cento dei cittadini italiani, secondo l'ultimo sondaggio, sono favorevoli alle dimissioni del presidente Renzi. presidente Renzi. Lo Stato italiano e i cittadini italiani stanno chiedendo al presidente Renzi di dimettersi. Ahimè, Renzi non lo fa e di conseguenza noi siamo costretti a chiedere le dimissioni con una mozione di sfiducia a questo Governo.

chi è da una parte e chi, come al solito, è dall'altra e appoggia come sempre questo Governo; un Governo che non avrebbe i numeri, ma che, come al solito, è appoggiato dai soliti noti eletti nelle fila di chi sta da questa parte e che, per una scelta di "cadrega", è ancora una volta dall'altra parte. Devono essere chiare le cose, in modo che i senatori e gli onorevoli del Partito Democratico la smettano di andare in televisione a dire che il signor Verdini non li sta appoggiando. Ancora oggi andavano in televisione e in giro a dire:

Presidente, qualcuno ci accusa di eccesso seriale di richiesta di sfiducia. Il problema non è questo, ma il fatto che c'è un eccesso seriale di richieste di fiducia da parte della maggioranza sui provvedimenti del Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).* Ciò che è irrituale in quest'Aula è la sequenza di richieste di voti di fiducia sui provvedimenti che la maggioranza dovrebbe essere in grado di approvare da sola, trattandosi di una forte maggioranza, e non dovendo avere teoricamente bisogno ogni volta di un voto di fiducia. La richiesta di voto di sfiducia che noi abbiamo avanzato è lo strumento parlamentare classico e tipico per approfondire un particolare argomento, che in questo caso è particolarmente complesso. È complesso non per lo scandalo, tutto da verificare, non per il Governo da mandare a casa, ma per quello che leggiamo nelle prime, cinque, sei, sette pagine dei quotidiani nazionali di tutti i giorni che riguardano membri del Governo.

quando in esse non c'è notizia di reato, ma quando vediamo un Ministro in carica (allora era ancora in carica) che, piangendo, colpevolizza il proprio compagno di vita di atti e fatti che riguardano però la sua attività di Governo, c'è un complesso di informazioni che hanno attinenza con l'attività di Governo su argomenti particolarmente importanti e sui quali - lo dico alla maggioranza - mi sembra più consono a questo Parlamento un dibattito in quest'Aula. Oppure lasciateci la possibilità di andare su tutti i *media* a dire le cose peggiori dell'Italia, del Paese, del Governo, della maggioranza, di esponenti politici, senza avere mai un momento di sintesi in cui questi argomenti possono essere affrontati con rigore, serietà e anche approfondimento reale e concreto (perché in Parlamento, teoricamente, le bugie non si dovrebbero dire). Questo è il motivo per cui abbiamo scritto una mozione di sfiducia, con la Lega in questo caso, e il motivo per cui abbiamo chiesto questo dibattito. Penso che sia interesse del Governo e della maggioranza che questo dibattito venga affrontato. Certo che può avere un minimo di attinenza con il *referendum* del 17 aprile.

*onshore*), e quale sia la politica del Governo in campo energetico (perché anche di questo si parla e di questo si è parlato) può essere un argomento interessante, visto che i cittadini italiani si trovano a dover votare - se intendono farlo - il 17 aprile. Quindi ci sembrava di capire e di fare una proposta che fosse concreta, reale ed in linea con le premesse che ho fatto, sulla quale pensavo che la maggioranza avrebbe deciso per il meglio; invece ha voluto in ogni caso e comunque posporre. Il problema non è la 17 aprile, ma è che da oggi al 19 aprile passeremo tredici giorni a leggere ancora una volta i giornali per sapere cosa sia effettivamente successo su problematiche molto, molto rilevanti. Prenderemo atto di quello che verrà scritto sui giornali e leggeremo sicuramente altre intercettazioni (perché mi pare che ne siano in arrivo altre), ma non sapremo qual è la posizione del Governo. Questa mozione di sfiducia era l'occasione perché questo dibattito avvenisse in questa sede, con il rigore che è tipico tipico di quest'Aula. Spiace che la maggioranza non abbia voluto avere questo coraggio. Ribadisco la mia richiesta, che ho già avanzato in Conferenza dei Capigruppo, che questa mozione di sfiducia venga analizzata e dibattuta martedì prossimo, martedì prossimo, all'inizio della settimana prossima, perché ritengo che questo sia un atto dovuto per rispetto a noi, innanzitutto, ed anche al Paese.

essa deputato. Peraltro non si è dimessa per motivi personali, ma si è dimessa per dei fatti ben precisi. Quindi trovo veramente grave, molto grave,

lo dico anche al collega Romani - non è vero che la questione e l'oggetto del *referendum* non c'entrano con quello che sta accadendo e con gli elementi che stanno emergendo giorno dopo giorno, in continuazione, dall'inchiesta e che noi evidentemente possiamo solo leggere e commentare sui sui giornali, ma non affrontare qui, nel luogo deputato. Il *referendum* c'entra eccome, perché il quesito referendario, quello sopravvissuto, riguarda quello che io ritengo un altro regalo alle solite società petrolifere, perché mantenere in vita le concessioni, fino a fine vita, significa fare un regalo alle società petrolifere. Quando vi è un'inchiesta ed emergono elementi di un sistema - come lo vogliamo chiamare? Un sistema di educande? - che coinvolge il livello locale e il livello dei Ministeri, per le cose continue che stanno emergendo, ancora non si vuole affrontare qui le cose per come sono? I cittadini prima di andare a votare debbono o no sapere se questo Governo persegue l'interesse generale o se, invece, persegue soltanto gli interessi di pochi? È una È una questione che meritava o no di essere discussa, nel momento in cui si stanno affrontando - la prossima settimana - gli ultimi giorni di campagna elettorale? Non debbono forse i cittadini avere tutti gli elementi? Se la maggioranza ha questi elementi e può chiarire che ha lavorato, che le scelte strategiche dal punto di vista energetico sono state fatte nell'interesse dei cittadini, venga qui, affronti la discussione. Abbiamo il diritto o no

Come mai, visto che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare con spirito di innovazione per il futuro del Paese? Questo abbiamo chiesto. Credo, signor Presidente, che vi sia un problema di dignità di questo Parlamento. Non si è mai visto che, dopo quello che sta emergendo, la maggioranza, ancora una volta, si sottragga e tenti di spostare e di dilazionare il confronto nel tempo. - lo dico con chiarezza - non pensiate che dopo il 17 aprile le cose saranno migliori. Probabilmente il 17 aprile i cittadini sapranno bene cosa votare e vi daranno un segnale chiaro e preciso, anche per tutto quello che sta emergendo. Chiediamo,

in modo serio - per quale motivo non sono stati fatti i monitoraggi ambientali nella terra della Basilicata; per quale motivo vengono costantemente ignorate tutte le prescrizioni minime; per quale motivo è stato perpetrato quello che noi riteniamo un vero e proprio attentato a

Signor Presidente, recita un adagio latino: *quieta non movere*. Credo che sia, forse, il dogma al quale questa maggioranza vuole piegare il dibattito parlamentare; ma credo anche che occorra fare delle riflessioni e l'Assemblea dovrebbe stare un po' più attenta a ciò che sta succedendo nel nostro Paese. I fatti della Basilicata, infatti, sono una spia rossa sul sistema democratico del Paese.

e preferisca fare un faccia a faccia in una televisione ormai completamente prona alla propaganda del sistema ci sta tutto. la plutocrazia che avanza, ossia tutti questi sistemi forti che continuano a spingere sotto il peso

Ci sono fatti che possono tranquillamente essere raccontati. Non si agitino i colleghi del Partito Democratico, perché quando ci sarà data la possibilità di discutere

Il gioco sporco su cui insiste questo sistema è continuare a tenere i cittadini in uno stato di bisogno, per cui il Presidente del Consiglio può andare in televisione a dire coloro che sono contro lo sviluppo non vogliono i posti di lavoro. Se i posti di lavoro devono essere contrabbandati affinché i cittadini delle nostre Regioni non possano essere nelle condizioni di veder garantito il minimo sindacale delle loro condizioni sanitarie e fisiche, ciò vuol dire continuare a rubare, non solo il lavoro, ma anche la salute dei cittadini italiani. Sulle questioni della Basilicata, c'è un dato fondamentale che dovrebbe emergere dal dibattito e che racconteremo; vorrei però capire se è possibile farlo nei tempi dovuti, oppure dobbiamo aspettare il giochino che sottende questo spostamento.

è che, con questo risultato referendario, il Presidente del Consiglio vorrebbe seppellire anche il *referendum* del prossimo autunno. Stia però tranquillo, perché quella battaglia la faremo fino in fondo. se, con le cose che la magistratura andrà a scoprire, alla data del prossimo *referendum* egli sarà ancora Presidente del Consiglio.

19 aprile - e portarsi a casa una riforma costituzionale con una maggioranza asservita, che tutto sa fare tranne che la cosa giusta per questo Paese.

La riforma costituzionale dovrebbe inoltre portare la firma dei veri Padri costituenti e non di quelli che si sta inventando! Siete vergognosi. Lei, Presidente del Senato, della Camera alta, sta permettendo che un Governo che non sa nemmeno se in questa Camera ha la fiducia, nell'altro si porti a casa la riforma costituzionale. Vergognatevi! E lo anticipi, anche domenica!

però l'impressione che, ormai ripetutamente in quest'Assemblea, viene praticato uno sport di grande esercizio di mandibole, lingue, narici e trombe di Eustachio, L'unico organo che non viene utilizzato è il nostro sistema cerebrale

Credo che proporre di discutere ulteriormente la fiducia a questo Governo sia assolutamente legittimo, siccome abbiamo la scadenza del 17 aprile per un *referendum* su questioni precise e specifiche, chiedo che sia sospesa l'attività d'Aula della prossima settimana, perché voglio discutere con i cittadini italiani del senatore Crimi)*. È necessario sollevare quel velo di ipocrisia e di nebbia che c'è su queste questioni. Pertanto, non credo che dobbiamo venire ad allenare le nostre mandibole, le nostre lingue e narici

il senatore Buemi continua a dire che non bisogna utilizzare la lingua, le trombe di Eustachio e chi più ne ha più ne metta, ma, nel momento in cui il senatore Buemi insulta i senatori che hanno presentato le mozioni di sfiducia dicendo che non utilizzano il cervello, consiglio al senatore Buemi di utilizzare la lingua

M5S).* Faccia le sue valutazioni politiche, ma evitiamo di esasperare e strumentalizzare ulteriormente

Ed è altrettanto evidente che il Governo non vuole che si svolga prima il dibattito perché ha paura che possano emergere degli elementi che guastano la festa al manovratore, il quale, nel frattempo, ha messo in atto una serie di manovre diversive che non ci stanno sfuggendo. L'uscita degli 80 euro ai pensionati fatta adesso, potuto farla uno o due anni fa. Se 3 miliardi di euro di debito si possono fare adesso, potevano essere fatti anche prima, salvo che a lui non interessi sollevare i pensionati indigenti dalla loro situazione di povertà, ma interessi esclusivamente mettere un diversivo sul tavolo per deviare

tutto. Questo è quello che ha intenzione di fare. Ebbene, signor Presidente, il dibattito nel Paese è oltre la maturità e mi preoccupano molto gli scontri di oggi a Napoli, perché era da tempo che non si vedevano le piazze infiammarsi quando arriva il Presidente del Consiglio dei ministri. Oggi a Napoli è successo anche questo.

per compiacere un Presidente del Consiglio dei ministri che manda il Ministro per i rapporti con il Parlamento in televisione a paragonare il dibattito sulla sfiducia a una partita di calcio. Mi domando se sia questa la serietà che contraddistingue il Governo. *(Applausi

Questo non è un modo serio di governare, ma è un modo di ingannare i cittadini. *(Commenti* *dal Gruppo PD)*. Ricordi come ha iniziato il suo Ministero, il presidente Renzi, pugnalando alle spalle chi lo ha preceduto e stia sereno, perché i cittadini non dimenticano queste cose. Vergogna!

Visto che ci avete fatto il "pacco" dell'emendamento e il "doppio pacco" di far discutere della mozione di sfiducia due giorni dopo il *referendum*, vi chiedo di fare un "contropaccotto" e di discuterla due giorni prima, cioè venerdì.

forse veramente è il caso che il Governo se ne vada a casa. E perciò, con più forza e a maggior ragione, noi chiediamo che venga discussa la mozione di sfiducia.

Signor Presidente, con gli ultimi fatta di cronaca il Governo si è messo obiettivamente in difficoltà. Correttamente le opposizioni stanno chiedendo un momento di chiarimento politico che ci è dovuto: è dovuto a noi come opposizioni ed è dovuto al popolo italiano perché si chiarisca le idee. il nesso tra questi fatti, che sono all'origine delle difficoltà del Governo, e il *referendum* del giorno 17,

Quindi, per il Governo, laddove abbia delle buone motivazioni e delle buone argomentazioni da addurre, sarebbe conveniente presentarsi in Aula e difendersi a testa alta di fronte all'opposizione. È utile, anzi necessario, per gli italiani capire chi li governa, come li governa, e capire perché loro di non andare a votare in un atto assolutamente nobile come quello dell'espletamento della democrazia diretta su un tema che li interessa.

si possa discutere la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni e dare così al Governo l'opportunità di difendersi nel luogo deputato. Ciò affinché in questo Senato, che è ancora un organo costituzionale ed è ancora la Camera alta di questo Paese, si possa trattare di politica, fare accuse politiche e difendersi in modo politico: qui in Senato, qui in Parlamento, e non in televisione, dove i giornalisti dimenticano di fare la famosa seconda domanda, quella che verifica la qualità della risposta data dall'intervistato.

Io non sono sorpreso da quanto sta emergendo sui giornali. E lo dico proprio a lei, signor Presidente, che so essere molto attento a questi problemi. Più volte ho denunciato che in tante Commissioni - fortunatamente non in tutte non si discute realmente di quello che viene proposto; gli emendamenti si discutono da altre parti. Più volte l'ho detto, quindi non sono sorpreso che alcuni emendamenti si discutano per telefono.

Presidente, credo che stiamo dando un cattivissimo esempio al popolo italiano, che sa bene quali esempi seguire e quali no. Soprattutto, stiamo scoraggiando un'intera Nazione rispetto alla possibilità di vedere i propri diritti e la democrazia tutelati dentro queste Aule.

Eugenio Cefis, che fu vice presidente e poi presidente dell'ENI dal 1967. Agli allievi cadetti in quell'occasione pronunciò parole terribili. Ne riporto alcuni estratti perché veramente sono di attualità e ci dicono quanto noi stiamo perdendo, giorno giorno dopo giorno, anno dopo anno, in termini di sovranità e quanto i poteri forti già avevano deciso della riduzione della sovranità popolare: il tradimento dell'articolo 1 della Costituzione. A pagina 8 di quel testo si legge: «Anche nelle decisioni di investimento le imprese hanno attribuito un'importanza secondaria ai confini nazionali, scegliendo per i nuovi impianti la località che poteva apparire più proficua, indipendentemente dal fatto che

oltre due terzi della produzione industriale mondiale sarà in mano alle 200/300 maggiori società multinazionali». A pagina 11: «Fino a quando il nostro Continente sarà frammentato in diversi Stati, fino a quando la multinazionalità potrà essere identificata con uno o due Paesi d'origine, cioè con i Paesi delle società madri, le iniziative delle affiliate della multinazionale dovranno sempre combattere un certo clima di diffidenza». «al limite può accadere talvolta che qualche Governo proceda alla nazionalizzazione di singole unità produttive appartenenti alla multinazionale. Ma è difficile che un tale Governo riesca a reggere alla pressione politica che le multinazionali possono esercitare». si dice: «è molto difficile che un Paese ancora povero e arretrato possa permettersi di adottare iniziative politiche che scoraggino gli investimenti esteri. Le *royalties* che vengono versate al Paese ospitante,» - ancora non si parlava di mazzette «la valuta derivata dalle esportazioni, i salari con cui la manodopera locale è retribuita, sono fatti economici di tale rilevanza da porre in secondo piano i problemi dell'autonomia e del prestigio politico». pagina 15: «ci si evolve sempre più verso l'identificazione della politica con la politica economica». E ancora: «se i controlli statali creano vincoli eccessivi agli investimenti e alle operazioni in un Paese, la società multinazionale può comunque agire potenziando le sue attività

che minaccerebbe 11.000 posti di lavoro. Questi sono i ricatti a cui dobbiamo continuamente sottostare sul piano mediatico. E abbiamo avuto dalla magistratura in questi giorni

del paravento sull'ipocrisia del Governo, noi non possiamo andarcene a casa. Io chiedo che il calendario sia cambiato e non ci si muova più da quest'Aula finché sul Governo Renzi non si sarà potuta discutere la mozione di sfiducia, altrimenti stiamo prendendo in giro gli italiani, seguendo un copione già scritto decenni fa, stiamo seguendo una manfrina che svuota completamente queste Aule di significato, stiamo perdendo il senso della nostra presenza qui dentro. Io spero, Presidente, che lei abbia orgoglio del senso della sua.

Presidente, ho chiesto di intervenire per annunciare a lei e all'Assemblea che ho scritto, insieme ai colleghi Guerra, Albano, Migliavacca, Rossi, Cuomo e Puppato, al presidente della Commissione di vigilanza RAI, onorevole Fico, una lettera di protesta contro Bruno Vespa. La trasmissione «Porta a Porta» è sempre stata la patria del *trash*, ma oggi abbiamo passato il segno: oggi siamo al salotto televisivo dove la mafia è di casa. Ad agosto 2015 Bruno Vespa ospitò i Casamonica e i loro avvocati; ne seguì una polemica e l'audizione del direttore Leone in Commissione d'inchiesta antimafia. In quella sede chiesi un procedimento disciplinare contro Bruno Vespa. Evidentemente non accadde nulla, quindi Vespa si è permesso di invitare Riina. Se potesse, inviterebbe anche Matteo Messina Denaro;

Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, tutti gli agenti delle loro scorte, e tutte le vittime della mafia che sono l'Italia migliore che Vespa non conosce, perché non la capisce. Vespa non aiuta i telespettatori a conoscere le logiche e la mentalità della mafia; egli è il cerimoniere del salotto della mafia. [**Presidenza del vice

certifica che esiste uno Stato e un anti-Stato. Signor Presidente, a tanto non si era mai arrivati. Chiedo le dimissioni dell'intero gruppo dirigente della RAI e del ciambelliere Vespa *(Commenti dal

che ogni giorno lottano con la

praticare la pacatezza, ricordo storicamente che il nostro collega Sergio Zavoli, che è un grande giornalista, intervistò per la televisione pubblica il terrorista Moretti, l'assassino di Aldo Moro, un terrorista che non è mai dissociato dalla lotta armata. Ricordo inoltre che Santoro ha interrogato Ciancimino a proposito di mafia. Ritengo pericolose e fuorvianti, anche se posso concordare su alcune valutazioni, le censure preventive, quando nessuno ha ancora visto la trasmissione di questa sera

collusione con le Brigate Rosse, perché ha intervistato il brigatista Moretti, che è pur sempre stato l'assassino di Aldo Moro. Detto questo, anch'io oggi ho detto che sono a disagio davanti a questa trasmissione

per attività mafiosa. Però detto questo, colleghi, toni come questi di aggressione ad un giornalista e di censura preventiva vanno bene nei Paesi totalitari, ma non vanno bene nei Paesi democratici. invito tutti alla compostezza e magari a dare un giudizio sull'accaduto quando ci sarà stata data l'occasione, per chi lo vuole fare questa sera, di vedere com'è stata impostata l'intervista che Bruno Vespa farà al giovane Riina.

tutti trasversalmente molto, molto grave. In primo luogo perché abbiamo il precedente dei Casamonica, in cui non c'è stato un lavoro giornalistico, quanto piuttosto un lavoro di estetizzazione della mafia, cosa che ritroviamo anche nell'eventualità di stasera. Non solo, stasera abbiamo un pregiudicato, che ha scontato otto anni per associazione mafiosa, che ha scritto un libro su suo padre, un *boss* mafioso attualmente in carcere, e che va a promuovere il suo libro in uno spazio pubblico e con soldi pubblici.

Quindi tutto quello che si può fare è chiedere immediatamente - e questo la Commissione di vigilanza lo farà - la convocazione del direttore di RAI 1 in in vigilanza RAI già la settimana prossima. Siano avvertiti che stasera, sulla base di come andrà questa trasmissione, noi chiederemo le dimissioni *in primis* di Vespa, che deve smetterla di fare queste cose (siamo tutti stanchi), e poi vedremo anche di stabilire le altre responsabilità. Noi, come Movimento 5 Stelle, invitiamo i cittadini italiani a non guardarlo stasera, perché l'operazione di Vespa è vergognosamente un'operazione di *share*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Voglio anche ringraziare il presidente Grasso, che oggi ha dichiarato che lui non la guarderà. Invito quindi tutti i cittadini italiani a fare la stessa cosa.

Non farei delle battaglie e non mi assocerei a quanto sostenuto dal collega Giovanardi, perché il tentativo non è quello di mettere la museruola ai giornalisti. L'aspetto scandaloso di quello che accadrà stasera a «Porta a Porta» è che, per poter fare spettacoli di questo genere (ormai tutto quanto fa spettacolo), queste cose vengano fatte con i soldi miei e dei contribuenti.

ma certamente c'è un tema che lei, in qualità di Presidente di questa seduta ma anche di commissario, come me ed altri, si dovrà porre. Il tema è che la vigilanza RAI

per insistere sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare che faccia chiarezza sulla ricostruzione *post* terremoto. L'Aquila non ha sicuramente bisogno di polemiche, bensì di provvedimenti concreti, che garantiscano trasparenza rispetto della legalità nella ricostruzione, per un territorio che è stato colpito da questo dramma. A noi di Italia dei Valori interessa questo; le polemiche le lascio volentieri agli altri.

ma devono lavorare per la ricerca della soluzione che sia il bene della popolazione, senza secondi fini e senza interessi personali. Questo equivale per me a sporcarsi le mani

ci sono momenti di commozione e commemorazione, c'è il minuto di silenzio, cui tutti si associano, ma dopo il minuto di silenzio, aprire un dibattito durante il quale la gente se ne va e chiacchiera, nel disinteresse generale, diventa anche indecoroso. quando una commemorazione diventa uno scontro politico, in cui vengono inseriti giudizi ingenerosi o di parte, assolutamente fuori luogo. Ho ritenuto di dover intervenire a fine seduta per dire queste cose, affinché anche a L'Aquila si sappia che nel Senato, in questa occasione, non c'è stata soltanto polemica politica.

ha ammesso centinaia di laureati sprovvisti di abilitazione. A questo provvedimento del giudice amministrativo seguiranno sicuramente ulteriori provvedimenti analoghi, con la conseguenza che anche soggetti sprovvisti di abilitazione all'insegnamento verranno ammessi alla procedura concorsuale, creando ulteriore confusione in un *iter* già abbastanza farraginoso. Quindi, caos su caos. pertanto se non sarebbe opportuno annullare il concorso bandito, proponendo eventualmente un altro concorso articolato in due fase conseguenti, che distinguano nettamente i soggetti non abilitati da quelli abilitati. Mi sembra abbastanza palese che questo concorso sia un raggiro: lo si vuole far passare per uno svuotamento delle graduatorie